senatori, prima di continuare con l'ordine dei lavori, consentitemi di rivolgere un affettuoso saluto di bentornato al presidente emerito Giorgio

Caro Presidente, credo che la sua capacità di partecipazione ai lavori e la sua passione istituzionale siano il miglior esempio per tutti i componenti di quest'Assemblea. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018 Dopo l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, avrà luogo la discussione, i cui tempi sono stati ripartiti fra i Gruppi per complessive

Signor Presidente, gentili senatrici, gentili senatori, il Consiglio europeo a cui parteciperò a Bruxelles, il secondo del Governo che presiedo, arriva in un momento in cui, anche rispetto a quello di giugno, è ancora più evidente in tutta l'Europa la viva aspettativa da parte dei cittadini di ricevere dalle istituzioni europee risposte e soluzioni concrete. Nell'agenda del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre e dell'Eurosummit del 18 ottobre sono inclusi temi cruciali quali l'immigrazione, la Brexit, il completamento dell'Unione bancaria. A questi temi si aggiungono quelli della sicurezza interna, che in parte abbiamo già trattato nel pre-vertice informale che si è svolto a Salisburgo il 19 e il 20 settembre, il capitolo delle relazioni esterne. Questo Consiglio europeo arriva in una fase particolarmente importante per il progetto europeo. È infatti iniziato il periodo conclusivo del cosiddetto ciclo istituzionale. Le elezioni europee, che sono fissate a maggio 2019, apriranno la strada alla designazione della nuova Commissione e del nuovo Presidente del Consiglio europeo. Soprattutto il percorso verso le elezioni europee vede l'Unione di fronte a quattro sfide, le cui risposte sono improcrastinabili nella stessa percezione dei cittadini europei. La prima sfida è quella di lavorare per una gestione condivisa multilivello dei flussi migratori, che consenta di affrontare un problema ormai di carattere globale con un cambio di paradigma - come noi abbiamo suggerito sin dall'inizio privilegiando un approccio strutturale a un approccio emergenziale, partendo dai movimenti primari per arrivare a quelli secondari. Occorre dare una risposta comune, con la definizione di un meccanismo stabile e sostenibile già nelle fasi di sbarco, redistribuzione e rimpatrio, senza oneri aggiuntivi per i Paesi come l'Italia di primo arrivo. Sono gli obiettivi di una regolamentazione efficiente e puntuale, inclusi nella nostra European Multilevel Strategy for Migration, con i quali l'Italia, grazie al suo significativo apporto, ha contribuito a invertire la tendenza in Europa dal Consiglio europeo di giugno. C'è poi il nodo della Brexit, che va sciolto arrivando a un accordo di recesso tra Regno Unito e Unione europea che tuteli i diritti acquisiti dei cittadini europei residenti nel Regno Unito, le relazioni economico-commerciali, per l'Italia in particolare le indicazioni geografiche e la sicurezza. Una terza sfida è quella della stabilità economico-finanziaria, della *governance* dell'Eurozona e del completamento dell'Unione bancaria europea. Per il nostro Paese è fondamentale ridurre il *gap* di crescita con l'Unione europea, orientando la politica fiscale di spesa pubblica a una prospettiva di crescita economica stabile e sostenibile. Al contempo, sosterremo la necessità di creare un vero meccanismo europeo di protezione dei depositi bancari, ovvero il terzo pilastro a compimento dell'Unione bancaria. L'impegno dell'Italia per il completamento dell'Unione economica e bancaria resta immutato. Il sistema Paese nel suo complesso si è adoperato per adottare importanti ed efficaci misure di riduzione del rischio del sistema bancario. Tra i vari progressi conseguiti segnalo che le sofferenze nette, cioè al netto delle svalutazioni e degli accantonamenti già effettuati dalle banche con le proprie risorse, a luglio 2018 erano pari a 40,1 miliardi, quindi quasi 26 miliardi in meno dei valori osservati un anno prima. Rispetto al livello massimo delle sofferenze nette, raggiunto a novembre 2015, pari a 88,8 miliardi, la riduzione è stata quindi significativa, di 48,7 miliardi. Oggi il rapporto tra sofferenze nette e impieghi totali si è ridotto al 2,3 per cento; era il 4,9 alla fine del 2016. quarta sfida è il negoziato per un nuovo e ambizioso bilancio europeo pluriennale, il quadro cosiddetto finanziario pluriennale, in cui chiederemo di spendere meglio le risorse destinate alla gestione dell'immigrazione; in più chiederemo maggiori risorse per sicurezza e crescita, ma certo non accetteremo che siano ridotti i contributi per l'agricoltura e la coesione. Nella prima interlocuzione sul prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027, ho già espresso la necessità di avere un'Europa più forte, più equa e più solidale, con un'attenzione particolare al problema della povertà e del divario territoriale, con un utilizzo sapiente dei fondi strutturali dedicati a questo tema; un'attenzione maggiore al lavoro, alla crescita, alla competitività, all'innovazione e all'inclusione sociale, tenendo al centro i nostri giovani con un contributo ulteriore al fondo sociale europeo; un bilancio dell'Unione moderno per affrontare le sfide comuni e sostenere la crescita nazionale. Lasciatemi cogliere questa occasione per sottolineare l'urgenza di un cambio di passo dell'Unione europea, che deve proiettarsi sempre più verso le esigenze della società civile, essere più vicina ai popoli e ai cittadini. L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione europea e un contributore netto al bilancio dell'Unione. Forti di questa nostra posizione, andiamo a Bruxelles con una manovra economica - come sapete - appena deliberata, di cui siamo orgogliosi e sulla quale intendiamo avviare un dialogo, confrontandoci senza pregiudizi. Siamo convinti che quella dell'*austerity* sia una strada non più percorribile. Tutte le misure al centro della manovra economica, sulla quale il Governo è impegnato e che certamente avrò modo di illustrare in maniera esaustiva anche alle istituzioni europee, ai nostri *partner* dell'Europa, sono improntate a favorire crescita, occupazione e a contrastare la povertà nel segno della stabilità sociale. Su questo posso garantirvi che il Governo tutto sta lavorando con consapevolezza e responsabilità senza sosta. L'architrave della nostra manovra è costituito dagli investimenti, ossia la componente che è mancata maggiormente nelle politiche economiche degli ultimi anni, che hanno determinato un ritardo di crescita del nostro Paese rispetto alla media europea. Per rilanciare gli investimenti agiremo su tre fronti: risorse, semplificazione delle procedure e potenziamento delle competenze e delle capacità progettuali del sistema Paese. Gli anni della crescita economica ci hanno insegnato che una società con profonde disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza non è soltanto moralmente inaccettabile, ma rischia di frustrare e fare implodere l'economia stessa. Un Paese che ha 5 milioni di poveri ha un problema evidente di giustizia distributiva e di tenuta sociale. Perfino le istituzioni internazionali, come il Fondo monetario internazionale, sostengono da tempo che un Paese con forti diseguaglianze sociali ed economiche non può essere stabile. Lo stesso Fondo monetario internazionale nel 2017 chiedeva all'Italia di dotarsi di uno strumento universale di *welfare* e anche nel pilastro europeo dei diritti sociali viene ribadita la necessità di stabilire un programma di reddito minimo collegato al reinserimento nel mondo del lavoro. L'Italia rimane un attore indispensabile affinché le quattro sfide, che ho appena citato e riassunto, trovino una soluzione europea efficace e convincente. Questo ruolo intendiamo giocarlo con il massimo impegno, perché consideriamo l'appartenenza all'Europa parte irrinunciabile del programma di miglioramento delle condizioni socioeconomiche dei cittadini italiani e dei cittadini europei. Adesso permettetemi di entrare più specificamente nell'ordine del giorno delle varie questioni. In tema di immigrazione, nei lavori del Consiglio europeo si farà una prima valutazione sulle articolate conclusioni sottoscritte nel vertice dello scorso giugno. Abbiamo lavorato, e continuiamo a farlo, affinché nelle conclusioni di questo Consiglio europeo venga rispettata la priorità di un'equilibrata e tempestiva attuazione di tutti i contenuti che sono già passati nelle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso giugno. In sostanza, continuiamo a considerare irrinunciabile che Stati membri e istituzioni comunitarie siano coerenti con quel cambio di prospettiva. Abbiamo infatti ottenuto che l'approccio europeo alla gestione della migrazione vada in direzione di un indispensabile equilibrio fra movimenti primari e movimenti secondari, di un riconoscimento del principio degli sforzi condivisi per gestire i migranti a seguito di un salvataggio in mare. In questo Consiglio europeo è dunque essenziale riaffermare l'impegno dell'Unione europea a rafforzare la collaborazione con i Paesi di origine e di transito e a investire di più e meglio nella gestione dei movimenti primari. Riaffermerò dunque l'elevata priorità di un rifinanziamento consistente e tempestivo da parte degli altri Stati membri del Fondo fiduciario dell'Unione europea per l'Africa, tecnicamente il Trust Fund for Africa. Investire per l'Africa oltre che in Africa è una priorità che ho sottolineato anche nella recentissima visita in Etiopia ed Eritrea, lo scorso 11 e 12 ottobre. La stabilità politica in quell'area, resa di nuovo possibile grazie allo storico accordo di pace firmato tra i due Paesi - l'ultimo il 16 settembre è infatti essenziale e va incoraggiata offrendo una prospettiva socioeconomica che disincentivi sempre più il ricorso ai canali illegali della migrazione come fonte di guadagno. La pacificazione e lo sviluppo dell'intera regione del Corno d'Africa possono assicurare senz'altro condizioni di vita migliori alle popolazioni locali e contribuire a stabilizzare - come ho rappresentato anche ai *leader* dei due Paesi - il quadro dei rapporti internazionali e i flussi migratori. Durante la mia visita, in particolare ad Addis Abeba, ho anche incontrato i vertici dell'Unione africana ad essi ho chiesto esplicitamente di farsi mediatori per incrementare gli accordi sui rimpatri, che oggi si fanno a livello bilaterale, e di sostenere la strategia che stiamo coltivando in Europa per la regolazione e la gestione dei flussi. In questa prospettiva, ho invitato i vertici dell'Unione africana a partecipare alla Conferenza di Palermo sulla Libia, che - come avrete già saputo - si terrà il prossimo mese di novembre. In questa direzione occorre anche che il Consiglio europeo incoraggi quell'alleanza Africa - Europa che lo stesso presidente Junker ha evocato nel suo ultimo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo. I movimenti primari, in sostanza, rimangono prioritari per una gestione europea sostenibile e duratura dei flussi migratori e degli stessi movimenti secondari. Questo concetto continuerò a rimarcarlo e a ribadirlo con gli altri *leader* europei. Occorre, infatti, evitare - a mio avviso l'illusione che i Regolamenti, e in particolare quello di Dublino, che riguarda il sistema europeo di asilo, possano risolvere le forti criticità relative ai movimenti primari e alla protezione dei confini esterni. Quando esamineremo la parte di conclusioni relative al contrasto del traffico di esseri umani e riguardanti la riforma del sistema europeo comune di asilo, richiamerò come ho già fatto a giugno - il fondamentale principio dell'equa condivisione delle responsabilità, sancito dall'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Anche su questo dobbiamo consolidare quel cambio di paradigma paradigma raggiunto al Consiglio europeo dello scorso giugno. Finché non riceveremo concrete garanzie sull'avvio della preparazione di questo meccanismo, non accetteremo a scatola chiusa accelerazioni sui movimenti secondari. L'ho detto da subito ai *leader* europei che hanno più a cuore questa parte della regolamentazione riguardante i movimenti secondari. Mi riferisco, in particolare, alla riforma del sistema europeo comune di asilo, su cui continuiamo a ritenere essenziale una «logica di pacchetto», che leghi l'avanzamento di tutti e sette gli strumenti legislativi che lo compongono. Mi riferisco anche alla proposta della Commissione di una Guardia costiera e di frontiera europea che costerebbe 11,3 miliardi di euro. di euro. Quest'ultima proposta desta nel Governo qualche perplessità. Personalmente mi riservo di fare una valutazione sia per il suo impatto sulla sovranità nazionale sia per gli elevati costi. L'Italia, infatti, ha già fatto molto e quasi sempre da sola grazie all'eccezionale impegno delle donne e degli uomini - voglio qui ricordarlo e sottolinearlo - della Marina militare e della Guardia costiera. Il riconoscimento da parte dell'Europa vogliamo che avvenga nei fatti e non solo negli apprezzamenti che ci sono stati dispensati nel tempo, e anche di recente, per aver protetto da soli negli ultimi anni

Dobbiamo farci trovare preparati nella nuova stagione degli arrivi e continuare a operare per la stabilità e la sicurezza del Mediterraneo. In questa prospettiva si colloca anche il nostro forte sostegno al processo politico in corso in Libia, obiettivo cui dedichiamo la Conferenza già menzionata in Sicilia, che si svolgerà a Palermo il 12 e il 13 novembre. Siamo impegnati a far sedere intorno a un tavolo tutti gli attori coinvolti nella stabilizzazione del Paese a sostegno delle Nazioni Unite. Continueremo a lavorare affinché i risultati positivi nella riduzione degli sbarchi si consolidano in un approccio europeo multilivello che assicuri risposte strutturali, le uniche capaci di dare sicurezza ai nostri cittadini. Per quel che riguarda specificamente la Conferenza in Libia, non abbiamo la presunzione di ottenere la risoluzione di tutti i problemi invitando tutti i principali *stakeholder* a sedere intorno a un tavolo a Palermo, ma sicuramente l'Italia - come è nelle sue corde e tradizione - è disponibile a farsi promotrice di questo processo di pacificazione e di stabilizzazione nell'interesse dello stesso popolo libico. Sono, dunque, qui a chiedervi di darmi il vostro sostegno per fare avanzare a Bruxelles l'impegno intrapreso fin dall'avvio dell'attività di questo Governo. Passando al tema Brexit, Passando al tema Brexit, vorrei ricordare che il capo negoziatore dell'Unione europea Michel Barnier - l'ho incontrato a Roma lo scorso 8 ottobre interverrà al Consiglio europeo a 27 (in questo caso) per fare il punto sugli sviluppi e sulle difficoltà, che avrete letto anche sui giornali, degli ultimi giorni. I 27 Capi di Stato e di Governo valuteranno lo stato dell'arte del negoziato in vista della ripresa dei colloqui tra il Regno Unito e l'Unione europea e di un possibile accordo a novembre. Domenica scorsa, i negoziatori del Regno Unito e dell'Unione europea hanno preso atto dell'impossibilità, al momento, trovare un'intesa sulla questione irlandese. È un tema complesso, in cui le ipotesi tecniche per evitare in concreto una frontiera fisica tra le due Irlande si intrecciano con importanti questioni, come sapete, di principio. I tempi sono davvero strettissimi. Dovremo lavorare tutti con buon senso, senza cedere alle emozioni e a reazioni istintive, per evitare un fallimento dei negoziati che - dobbiamo riconoscerlo e dirlo - sarebbe un salto nel vuoto, con presumibile effetto negativo per imprese e cittadini. È invece nostro dovere assicurare un recesso ordinato, seconda modalità che siano chiare e garantiscano la protezione dei diritti acquisiti dai cittadini europei, nonché la stabilità economica e finanziaria per le imprese. L'intesa finale dovrà essere rispettosa della volontà del popolo britannico di lasciare l'Unione europea e dei principi fondamentali dell'Unione stessa. L'accordo sulla Brexit dovrà assicurare, anche in concreto, la tutela dei diritti acquisiti dai cittadini europei, tra cui i circa 700.000 italiani residenti nel Regno Unito, attraverso procedure semplici e rapide, con particolare attenzione alla protezione delle categorie più vulnerabili. Un altro tema centrale per l'Italia e per molti Paesi europei è la protezione delle indicazioni geografiche e delle regole di origine. Qualsiasi intesa con il Regno Unito - su questo sono stato molto chiaro con il rappresentante e il negoziatore dell'Unione europea Barnier dovrà preservare e valorizzare questo imprescindibile patrimonio di conoscenze, tradizioni e opportunità economiche. Una volta concordati i termini del recesso con un accordo che regoli anche la complessa questione del confine irlandese, potremo lavorare con il Governo britannico per costruire un futuro partenariato economico e di sicurezza, all'altezza dei profondi legami tra Londra e il resto del continente europeo. È questo il nostro obiettivo principale dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, che mi auguro avvenga in termini chiari e amichevoli, senza strappi. Soltanto in un clima di solida amicizia e reciproca fiducia potremo trovare nuove modalità di cooperazione e costruire una relazione economica e di sicurezza tra l'Unione europea e il Regno Unito all'altezza dei legami storici, culturali e politici tra Londra, l'Italia e il resto dell'Europa. Anche dopo Brexit il Regno Unito resterà un Paese europeo, con valori e sfide comuni a quelle degli Stati membri dell'Unione europea. Londra sarà ancora un attore fondamentale nell'economia globale e nell'architettura di sicurezza europea. Del resto, non potrebbe essere altrimenti per un Paese membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del G7 e della NATO. L'Italia continuerà quindi a lavorare per un partenariato basato sulla mobilità, affinché possano continuare i fruttuosi scambi economici tra i nostri cittadini, cittadini, per mantenere un elevato scambio dei commerci, e sulla sicurezza, per affrontare insieme in maniera più efficace le numerose sfide del nostro tempo. Passo al tema della sicurezza interna. Al Consiglio europeo approveremo delle conclusioni anche sul tema della sicurezza interna, sulla scia della discussione, già parzialmente anticipata nel corso del vertice informale a Salisburgo. Sul contrasto alle interferenze, anche *online*, nelle elezioni e sulle minacce ibride e *cyber*, condividiamo con i *partner* europei, a cominciare dal Regno Unito e dai Paesi bassi, la forte preoccupazione relativa alle recenti notizie di attacchi cibernetici. Rispetto ad essi, Rispetto ad essi, l'approccio italiano è ispirato alla promozione di piattaforme cooperative e mira a coniugare le esigenze di sicurezza e di protezione dei cittadini con il rispetto della democrazia e della libertà della rete. Riteniamo inoltre che abbiamo il dovere di rafforzare la resilienza, cioè la capacità di dotarsi, a livello nazionale ed europeo, di adeguati strumenti di prevenzione e resistenza rispetto ad eventuali attacchi *cyber*, ma anche la capacità di deterrenza verso tali attacchi, rispetto ai quali il problema dell'attribuzione, e quindi di eventuali misure sanzionatorie nei confronti dei sospetti responsabili, resta di grande complessità. Guardiamo Guardiamo con favore al fatto che il Consiglio europeo dia impulso anche all'*iter* di revisione del meccanismo europeo di protezione civile. L'Italia considera infatti essenziale un sistema coordinato ed efficace di risposte sia alle minacce nucleari, batteriologiche, radiologiche, chimiche, sia alle catastrofi naturali.

sarà questa una nuova occasione per stabilire, con i colleghi europei, come declinare coerentemente l'approccio che definisco a doppio binario - cioè, fermezza, ma coniugata al dialogo nei confronti di Mosca, che resta un attore ineludibile per la soluzione delle principali crisi internazionali. Ricordo a questo proposito che il 24 ottobre sarò a Mosca a incontrare Putin e, in occasione di questa mia visita, avrò modo di confrontarmi con lui su temi internazionali e di sicurezza. internazionali e di sicurezza. La politica europea nei rapporti con la Russia resta legata ai cinque princìpi concordati a 28 nel marzo 2016: le sanzioni fini a se stesse non fanno che danneggiare le nostre imprese, che invece questo Governo intende tutelare e sostenere, e la stessa società civile russa. In questo quadro - già a giugno scorso, a dire il vero - abbiamo espresso l'esigenza di dare grande attenzione a tale aspetto, anche attraverso programmi di supporto alle piccole e medie imprese. In questa prospettiva, come ribadirò ai colleghi europei, riteniamo si debba continuare a ragionare mantenendo, però, l'unitarietà della posizione dell'Unione europea nei rapporti con Mosca. Signor Presidente, gentili senatrici e cari senatori, questa è la posizione che intendo rappresentare in sede europea. Chiedo il vostro pieno sostegno, nella ferma convinzione che sia questa la strada giusta per portare anche in Europa quel cambiamento autentico che i cittadini del nostro Paese ci chiedono e si aspettano. Vi ringrazio per l'attenzione.

finestra"). È presente in tribuna una delegazione bicamerale del Parlamento indiano, guidata dal ministro di Stato per gli affari parlamentari e per le risorse idriche, signor Arjun Ram Meghwal.

*(PD)*. Signor Presidente, colleghi senatori, Presidente del Consiglio, ritengo necessario partire dagli esiti del Consiglio europeo del giugno scorso, che ha coinciso, peraltro, con il suo debutto sulla scena europea. Il ricordo di questo evento è caratterizzato da un principale elemento: la contraddizione, che è il risultato del rapporto tra i suoi commenti trionfalistici e la loro successiva demolizione colpo su colpo, emersa con la lettura ufficiale dei documenti di quell'incontro e di retroscena riportati da suoi omologhi, i quali restituiscono la cifra della imperizia della nostra rappresentanza in quel consesso internazionale. Quanto accaduto a fine giugno si iscrive però nel perimetro delle modalità che caratterizzano la vostra azione di Governo e infatti ha due facce: la prima risponde alla propaganda ed è sempre trionfalistica, la seconda invece riguarda la realtà ed è sempre uno smacco. Ricorda un po' le fiammanti distese di armamenti degli anni Trenta del nostro Paese, un vero trionfo di acciaio italico. In realtà, però poi era pessimo e rabberciato cartone. Quel Consiglio europeo di giugno, scevro del sabotaggio delle solite manine che voi vedete in ogni dove, non ha portato alcun miglioramento rispetto alla gestione condivisa dei migranti, come lei afferma, semmai, al contrario, un preoccupante passo indietro, se penso all'introduzione del principio della volontarietà che cancella i progressi ottenuti nel precedente Consiglio del giugno 2015. Ma non basta. È stato messo un ulteriore paletto, quello della unanimità dei 27 Stati membri, per la procedura di revisione del Regolamento di Dublino. Basterà quindi un solo Orban di turno a far saltare qualsiasi possibilità di modifica. Non mi solleva in tal senso ricordare a me stesso che proprio Lega e MoVimento 5 Stelle già nel novembre 2017 fecero ancora peggio - se posso dire - prima di Orban, avendo votato non a favore della proposta di revisione di quel regolamento e delle politiche relative al diritto di asilo. signor Presidente, è inutile nascondere che l'aspetta un tavolo non facile, perché quello di Strasburgo sarà un Consiglio carico di temi dirimenti per il futuro assetto dell'Unione, dove la finalità squisitamente politica di questo organismo rende ancora più necessaria la credibilità e la capacità di produrre in quel consesso un'efficace sintesi degli interessi del nostro Paese. Un consesso dove siamo chiamati ad essere responsabili e credibili e meno innovativi di come invece ha già voluto dimostrarsi il ministro Savona con il racconto della sua vicenda del milioncino abbondante di euro nei conti svizzeri. una credibilità che spero smetteremo presto di disperdere in quella che si rappresenta ormai come una vera e propria emorragia che si protrae da mesi. Non potete continuare a confondere la rumorosità delle nuove grida manzoniane, le grida di Salvini che vi garantiscono alta visibilità, con la perdita di credibilità che il nostro Paese sta patendo sotto tanti, troppi aspetti, quelli della reputazione economica, come raccolto dai giudizi di diversi organismi di ogni ordine e grado, dai previsori internazionali all'Ufficio parlamentare di bilancio, fino a quella squisitamente politica con l'uso di toni incendiari che non celano mai l'insulto a chiunque osi obbiettare nel merito. Signor presidente Conte, vorrei essere ancora più chiaro. La scelta politica in ambito europeo non può assumere come termine ultimo l'appiattimento su scelte opportunistiche orientate solo alla prossima campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo. Dico questo perché già nel giugno scorso questo Governo si è piegato in modo imbarazzante agli interessi del gruppo di Visegrad, che sono obiettivamente contro quelli italiani e le finalità dell'Unione.

In altre parole, state appoggiando i vostri sabotatori, i nostri sabotatori, come in una tipica sindrome di Stoccolma. E questo non solo in tema di migranti, ma anche in quello più grave e preoccupante che riguarda proprio la natura di questa Unione, che è democratica, basata sullo stato di diritto e sul rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo. L'Europa politica che oggi conosciamo e che non sempre ci piace, perché - come sappiamo bene - necessita di affinare procedure maggiormente democratiche, è costata carne e sangue agli europei, ceneri e macerie al nostro continente. In questo senso, anche la Brexit assume un tono e un valore che dobbiamo farci carico di gestire con il peso della storia e del suo insegnamento. Dobbiamo scongiurare una *hard* Brexit, non solo per le ripercussioni economiche che andrebbero a gravare *(Richiami del Presidente)* - mi Presidente, un minuto - su uno scenario di rallentamento della crescita mondiale, già di per sé preoccupante, ma per salvaguardare i diritti degli italiani presenti sul territorio inglese, dal punto di vista sociale, del lavoro e della salute. Sono infatti 3,5 milioni gli europei che vivono sul territorio inglese e, tra questi, oltre mezzo milione gli italiani. Dico questo perché se le trattative sulla Brexit sembrano aver trovato qualche convergenza sulle tematiche dei diritti, tante altre questioni rimangono ancora aperte e tutte da risolvere. Una di queste concerne il territorio irlandese, che tornerebbe ad essere terra di confine, oltre allo Stretto di Gibilterra, tra il Regno Unito e l'Europa, d'Irlanda che rimarrebbe sotto il cappello dell'Unione europea e un Irlanda del Nord che, al contrario, seguirebbe le sorti del Regno Unito. Nessuno vuole - spero nemmeno lei, presidente che in quelle zone si ravvivino conflittualità che oggi sembrano sopite e che presto invece potrebbero riaccendersi, sulla base dei negoziati su come si intenda dirimere la questione del confine

per i motivi che richiamavo, e dall'altra dall'esigenza di tutelare tutte le nostre aziende rispetto all'ingresso di prodotti extraeuropei, che proprio dall'Irlanda del Nord potrebbero trovare una comoda porta di accesso. Noi del Partito Democratico chiediamo a lei, presidente Conte, di portare avanti le trattative nel preminente interesse dei cittadini italiani e delle aziende del nostro Paese, superando quell'ambiguità che ha caratterizzato la vostra azione sin qui. Infine, signor Presidente, un pensiero sulla sicurezza e sulla lotta al terrorismo. La sicurezza dell'Unione europea va declinata sotto diversi aspetti, da quella fisica, interna e verso l'esterno dei confini dell'Europa... PRESIDENTE. Io non ho l'abitudine di interrompere, senatore Stefano, però la pregherei di rispettare i tempi, perché li ha abbondantemente superati, *(PD)*. Ho finito. ...a quella più labile e più facilmente permeabile che caratterizza la rete. Questo infatti è forse il fronte più scoperto e più complesso del nostro sistema democratico, dove viviamo una sorta di invasione verticale, giacché il terreno del confronto assume caratteri fino ai tempi della cronaca non pensati e non pensabili.

per un ravvedimento operoso da parte di questo Governo rispetto al suo atteggiamento verso l'Europa, soprattutto sul delicatissimo tema delle migrazioni e della sicurezza. Sarebbe opportuno in realtà un ravvedimento da comunicare all'Europa anche sulla manovra finanziaria, glielo dico con grande franchezza; il punto in questo caso, visto che lei vi ha accennato nel suo discorso, non è tanto quantificare la percentuale di *deficit* che il nostro Paese può produrre, a fronte di una complicata condizione strutturale, ma come utilizzare l'indebitamento. Le ultime notizie, ancora senza indicazioni di coperture, ci hanno restituito l'idea che avete scelto di usare la manovra per una sempre presente campagna elettorale piuttosto che per migliorare, attraverso investimenti utili e di prospettiva, le condizioni di crescita e di sviluppo del nostro Paese. Torniamo però all'ordine del giorno. Non possiamo dimenticare come le dichiarazioni del giugno scorso, quelle nelle quali parlavate di vittoria in sede europea, siano state totalmente ribaltate dalle conclusioni del Consiglio, che ora dovrà valutare quanto è stato fatto in questi mesi. Signor presidente Conte, ci piacerebbe molto che lei ricordasse ai suoi colleghi che il Parlamento europeo che il Parlamento europeo ha avanzato una proposta seria e di buon senso. Bisogna cambiare il Regolamento di Dublino e occorre farlo ora, rafforzando il principio di solidarietà e abolendo una volta e per sempre il principio del primo approdo, che ha avuto conseguenze durissime per il nostro Paese e per il dibattito politico in sede europea. Bisogna distribuire secondo quote predefinite i richiedenti asilo in tutti gli Stati membri e ridurre l'accesso ai fondi UE per gli Stati che non vi ottemperino. La strada che il suo Governo propone è, a nostro avviso, errata. Del resto, uno dei suoi Vice, che troppo spesso appare come l'uomo che le detta la linea (quando dovrebbe essere il contrario), è alleato politicamente con chi vuole alzare muri e filo spinato piuttosto che cambiare le regole dell'Unione per realizzarla compiutamente e su basi nuove. In queste settimane appare evidente la cifra del Governo Lega-5 Stelle: essere forti coi deboli, sostenere politiche di esclusione dei bambini figli di stranieri dalle mense scolastiche e dagli aiuti per i libri, smantellare un modello di integrazione come Riace, ed essere deboli, debolissimi con i forti tramite *flat tax* e condoni fiscali. Nella nostra risoluzione troverà elencate una serie di misure volte a gestire con umanità e intelligenza il fenomeno delle migrazioni. La più importante è l'apertura immediata di corridoi umanitari di accesso in Europa per garantire canali di accesso legali e controllati, attraverso i Paesi di transito, ai rifugiati che scappano da esecuzioni, da persecuzioni, da guerre e da conflitti, per mettere fine una volta per tutte alle stragi in mare e in terra, e quindi debellare il traffico di esseri umani, anche con visti e missioni umanitarie. L'altra misura è quella di sostenere una riforma finalizzata a creare un reale diritto di asilo europeo capace di superare il Regolamento di Dublino: proprio quella misura contro cui hanno votato i suoi compagni di Governo. Le aggiungo una considerazione. La legge Bossi-Fini è quanto di più criminogeno si possa immaginare. Se non avete intenzione di abrogarla, ripristinate almeno il decreto flussi per chi lavora, anche solo per la reale necessità di famiglie e imprese. D'altronde, è ormai chiaro che risolvere problemi complessi non fa parte del contratto di Governo; anzi, più si creano situazioni di disagio, più proverete a cavalcarle, e questo comportamento ha un nome: si chiama cinismo politico ed è quanto di più lontano da una cultura di Governo si possa immaginare. L'Italia le sta dimostrando con piccoli e grandi gesti che il nostro popolo è molto più attento, sensibile e solidale di quanto vorreste. Le raccolte fondi per i bambini di Lodi e per la encomiabile iniziativa della nave Mediterranea stanno abbattendo ogni precedente per quantità e rapidità di adesione. Chiamiamole con una forma che possiate comprendere: sono queste le soluzioni del popolo ai problemi che il Governo del cambiamento non ha alcuna intenzione di affrontare. Sui temi della sicurezza vi chiediamo, tra gli altri, impegni concreti per approfondire la revisione del quadro penale europeo in materia di terrorismo; misure volte a sottrarre alle organizzazioni criminali e terroristiche gli strumenti necessari alle loro attività, come l'accesso alle risorse finanziarie, alle armi, all'utilizzo di Internet e di documenti contraffatti, così come il miglioramento dei sistemi di scambio di informazioni tra autorità di contrasto, Polizia e magistratura penale, così come quelle di *intelligence* fra gli Stati membri. Infine, una seria lotta al riciclaggio e ai paradisi bancari e fiscali. Dispiace molto notare, signor Presidente del Consiglio, che quel decreto-legge che avete chiamato decreto Salvini (lo ricorda? Ha fatto le foto col cartello) e che vendete come decreto sicurezza otterrà esattamente l'effetto opposto. Del resto, è già una prassi per voi dare bei titoli a provvedimenti che non avranno effetti positivi sulla vita reale. Infine, sulle relazioni esterne dell'Unione, come non vedere che Stati Uniti e Russia si muovono nella stessa direzione? È casuale? Trump ha riesumato la pratica e la politica della destra neoconservatrice americana, quella più nazionalista, che durante il primo mandato di George Bush parlò apertamente di eurominaccia. Le tensioni politiche e commerciali alimentate da Trump nei confronti dell'Europa non possono che incontrare il favore di Mosca, incrociando così le mire storiche di affermazione e di una influenza russa sui Balcani e sugli Stati baltici. Per realizzare tutto ciò, occorre che l'Unione europea si scomponga e si dissolva ed è questo l'obiettivo comune a Trump e a Putin. Troppe dichiarazioni e azioni dei sostenitori del suo Governo esaltano entrambi e le loro politiche. Anche su questo il suo Governo ci appare su una strada sbagliata. Presidente Conte, ogni giorno qualche cittadina e cittadino in più si rende conto della pericolosa china di rabbia, frustrazione e razzismo che sta prendendo il nostro Paese. Auspichiamo, per convinzione politica, che lei non si lasci cullare dai sondaggi. Altri, prima di lei, hanno fatto lo stesso errore. Non sono riusciti a cogliere il malessere crescente e la storia li ha puniti. Non sarà sulle macerie che il vostro consenso potrà crescere. La invitiamo, quindi, a riflettere su questo mentre sarà in viaggio per rappresentare il nostro Paese al Consiglio europeo. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, l'Europa si trova di fronte ad uno dei cambiamenti più importanti della propria storia: l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Una decisione dolorosa, che avrà ripercussioni profonde, non soltanto per il Regno Unito, ma per tutta l'Unione europea. Il Regno Unito ricopre, infatti, un ruolo di primaria importanza per l'Europa da più punti di vista, ma soprattutto in ambito economico, con un volume d'affari di circa 650 miliardi di euro annui. Stessa cosa per l'Italia, per la quale il Regno Unito rappresenta il terzo Paese di esportazione, con circa 23 miliardi di entrate ogni anno. Un indotto importante. Cambiamenti tra i due Paesi possono avere anche ricadute occupazionali gravi. che in queste settimane, a poca distanza dalla *deadline* per la conclusione degli accordi, sarebbe importante un contributo fattivo, anche da parte italiana. Invece, in questa importante discussione sulla Brexit, la più rilevante degli ultimi sessant'anni in Europa, la voce italiana non c'è stata. Assente, non pervenuta. È il segno che, neanche a cinque mesi dal suo insediamento, presidente Conte, l'Italia in Europa è isolata e gode di pochissima credibilità. Nella discussione sulla Brexit il Governo giallo-verde sembra dimenticarsi anche degli oltre 700.000 italiani che vivono e lavorano nel Regno Unito e che sono interessati personalmente dalle ricadute *post* Brexit. Italiani destinati a sperimentare sulla propria pelle gli effetti della riuscita o no dell'accordo tra Unione europea e Regno Unito. In questo processo è in ballo anche il loro futuro, la loro vita e quella dei loro cari, perché ne va del loro *status* di cittadini, di lavoratori, di studenti. Per noi del Partito Democratico è chiaro, è sempre stata la nostra linea politica. Va garantito il mantenimento di tutti i diritti conseguiti ai cittadini comunitari presenti nel Regno Unito, sia in ambito lavorativo che formativo, in campo sanitario, in ambito politico, nel settore universitario e della ricerca, nella vita quotidiana. Ma qual è la linea del suo Governo, presidente Conte? L'impressione è che, al di là delle rassicurazioni odierne, questi italiani le interessino ben poco. Al contrario, bisognerebbe garantire loro certezze, creando al contempo le condizioni per permettere un'uscita del Regno Unito dall'Europa il meno traumatica possibile. Un accordo potrà avere successo solo se va incontro a tutte le parti in causa. Al tempo stesso, è chiaro che non potranno essere concessi al Regno Unito gli stessi privilegi di cui godeva prima. Dall'evolversi dei fatti delle ultime ore, sembra non si riesca a raggiungere un accordo, il che potrebbe creare conseguenze negative. Ciò nonostante, credo non sia il caso che l'Europa adesso ceda alle pressioni solo per il timore delle conseguenze, perché non è affatto chiaro come saranno i prossimi sviluppi della politica interna britannica, già molto turbolenta nelle ultime settimane; anzi, non è escluso che arrivino altri al Governo, con la possibilità di scenari politici del tutto nuovi e magari anche un esito diverso rispetto alla questione Brexit. Brexit. Oggi, con il suo intervento, ha fatto capire che sulle politiche europee a lei e al suo Governo manca la bussola, perché fare promesse e sparare offese su Twitter, come sono soliti fare i suoi ministri, senza essere in grado di farsi ascoltare a Bruxelles nelle sedi che contano o senza presentarsi affatto - com'è successo ad esempio la settimana scorsa, e non era la prima volta - è proprio il contrario di una politica seria ed efficace; dunque è inevitabile poi tornare a casa a mani vuote.

perché non solo non ha conseguito risultati oggettivi, ma addirittura ha lasciato fare passi indietro madornali rispetto a quanto avevamo faticosamente conquistato con i nostri Governi:

adesso si potrebbe sanare solo attraverso una modifica del Trattato di Dublino, nella forma a suo tempo indicata dai nostri Governi, ribadita dal voto del Parlamento europeo. Bisogna superare il concetto di Paese di primo arrivo: i migranti vanno ripartiti su tutti i Paesi europei. Questa è la nostra proposta, una soluzione che aiuterebbe di fatto l'Italia:

questo Consiglio, di conseguire risultati a beneficio dell'Italia e degli italiani. Noi del Partito Democratico siamo molto preoccupati dell'evolversi del suo agire. Vediamo come sia crollata la capacità negoziale dell'Italia in Europa,

ci occupiamo di temi molto delicati e sentiti, lungamente dibattuti negli ultimi mesi e anni, che spesso hanno provocato contrapposizioni ideologiche, a volte strumentali alla lotta politica domestica. Il tema della pressione migratoria è stato affrontato dall'Unione europea probabilmente in modo tardivo e solo dopo la crisi del 2015. Da allora, sono state adottate una serie di misure che hanno sì ridotto complessivamente i flussi e controllato meglio le frontiere esterne, ma tali misure non sono state applicate in modo omogeneo, né era possibile farlo, considerata la diversità fisica tra le diverse frontiere dell'Unione europea, e ciò ha creato una pressione maggiore su alcuni Paesi, tra cui il nostro, e minore su altri. L'Unione europea ha più volte affermato che intende proseguire su questa politica del maggior controllo delle frontiere esterne ai fini del contenimento della immigrazione illegale su tutte le rotte, quindi sia su quella del Mediterraneo orientale e occidentale, sia su quella del Mediterraneo centrale, che è quella che ci riguarda più da vicino e che al momento crea maggiori preoccupazioni. Per disincentivare il traffico di essere umani nel Sahel, in Libia, nel Corno d'Africa e nel resto del continente africano, l'Unione europea deve sostenere le attività della Guardia costiera libica, a cui il nostro Paese ha donato motovedette proprio a questo scopo, favorire i rimpatri umanitari volontari, ma soprattutto deve cercare di eliminare o limitare i motivi che originano le migrazioni di massa, ossia i conflitti, la povertà, le diseguaglianze economiche e sociali. Questi obiettivi, come si vede, sono ambiziosi e radicali, perché si tratterebbe di favorire da un lato la composizione o cessazione di conflitti decennali, alcuni dei quali nati per lo sfruttamento di risorse naturali, e dall'altro si tratterebbe di intraprendere politiche di cooperazione volte alla trasformazione socio-economica del continente africano, sulla base dei princìpi e degli obiettivi definiti dalle Nazioni africane nella loro agenda 2063, nei settori nevralgici dell'istruzione, della salute, delle infrastrutture, dell'innovazione, del buon governo e della emancipazione femminile. Sono progetti ambiziosi, che presuppongono il significativo incremento delle politiche di cooperazione in termini di quantità e di qualità e di conseguenza saranno necessari maggiori fondi, ma anche misure intese a creare le condizioni che facilitino l'aumento degli investimenti privati, siano essi africani o europei. In conseguenza di tutto ciò, aumenteranno gli scambi commerciali tra Africa e Europa. Progetti ambiziosi, che noi tutti speriamo prendano corpo il prima possibile e che portino frutti nel più breve lasso di tempo, ma purtroppo, nell'attesa che tutto ciò accada (tra l'altro sento parlare di queste cose da quando ero ragazzo) occorre occuparsi di vite umane in pericolo sia in mare, sia nel deserto, sia nei campi in Libia, sia nel resto dell'Africa. Da questo punto di vista, l'Unione europea doveva e deve fare molto di più e invece spesso si è limitata a denunciare norme di principio, a tratteggiare programmi futuristici che però hanno lasciato alcuni Paesi più di altri sottoposti alla pressione migratoria, costretti a causa della loro posizione geografica a dover gestire l'accoglienza di centinaia di migliaia di esseri umani, di nostri fratelli bisognosi di cure. Per non scontentare i Paesi meno propensi all'accoglienza, l'Unione europea ha recentemente lasciato agli Stati membri la possibilità, su base volontaria purtroppo, di partecipare a un programma comune secondo cui chi viene salvato a norma del diritto internazionale dovrebbe essere trasferito in appositi centri da istituire in tutti gli Stati membri partecipanti, dove dopo una rapida attività di indagine dovrebbe essere possibile questo negli auspici - distinguere i migranti irregolari, che devono essere subito rimpatriati, dalle persone bisognose di protezione internazionale o di asilo, a cui si applicherebbe il principio di solidarietà. Se però la partecipazione a questi programmi non è obbligatoria e se non si modifica il regolamento di Dublino, la solidarietà europea rimane più sulla carta che nei fatti e di conseguenza l'accoglienza viene effettuata in gran parte da alcuni Paesi, tra cui il nostro, e poco o pochissimo o nulla A parole, le nostre frontiere esterne a Sud sono frontiere europee, ma nei fatti, o almeno fino ad oggi, sono frontiere italiane e tocca a noi gestirle, con tutto ciò che consegue in termini di costi economici e sociali. D'altro canto, le sofferenze e i soprusi cui sono sottoposti molti migranti sono per noi inaccettabili, perché cozzano contro i principi europei, con quelli della solidarietà e con la nostra dignità di uomini e donne. Considerato che siamo uno dei Paesi fondatori della Comunità prima e poi dell'Unione europea deve essere un nostro precipuo compito fare in modo che questa tendenza sia invertita e che quindi tutti gli Stati dell'Unione siano coinvolti nella gestione delle frontiere dei flussi migratori. Tutti, nessuno escluso. Non si può essere europei ed europeisti quando si devono ricevere i fondi e poi diventare nazionalisti quando invece si deve dare una mano ad un altro Paese europeo e ad essere umani che sono nostri fratelli e sorelle. Purtroppo molti errori sono stati fatti in passato e alcuni si ripetono ancora oggi. Mi riferisco, per esempio, all'intervento militare in Libia del 2011 che ha destabilizzato quel Paese, cui purtroppo partecipò anche l'Italia, o alle modalità di sfruttamento delle risorse africane da parte di alcuni Paesi europei, che si comportano non come *partner* commerciali ma quasi come se esistessero ancora le colonie, a volte tentando di condizionarne lo sviluppo socio-economico e causando vaste sacche di povertà; ciò è una delle concause all'origine dei flussi migratori. Il discorso sarebbe lungo e quindi torno alle attuali politiche europee in tema di immigrazione e sicurezza interna: criticarle non vuol dire essere euroscettici o peggio antieuropeisti. Proporre la revisione di trattati o regolamenti, cercare di riscriverli tenendo conto di quanto accaduto negli ultimi anni, sia di positivo e sia di negativo, non significa volere la fine dell'Unione europea. Il MoVimento 5 Stelle non è antieuropeista; al contrario, noi vogliamo rafforzare l'Unione, renderla più coesa, più giusta e più equa. Non vogliamo tornare indietro; al contrario, vogliamo andare avanti, vogliamo cambiare in meglio le cose. Tutto questo sta per succedere; le prossime elezioni del Parlamento europeo porteranno uno stravolgimento dell'attuale situazione politica e quello che è successo in Germania negli ultimi giorni è solo un prologo. Sapete, è ben strano sentirsi tacciare di antieuropeismo per il solo fatto di contrastare politiche europee rivelatesi profondamente sbagliate e questo accade sia nel campo della gestione dei flussi migratori sia, ad esempio, per ciò che riguarda il campo economico. Non si è antieuropeisti se si vogliono migliorare le cose; sarebbe come dire che chi è contro l'attuale Governo italiano è contro la forma repubblicana o che chi voleva cambiare la nostra Costituzione voleva distruggere lo Stato repubblicano e tornare alla monarchia. Sarebbero e sono concetti risibili, ma quando si parla di Europa ce li propinano come se fossero verità inoppugnabili. È vero l'esatto contrario; chi critica alcune scelte, chi vuole cambiare politiche, si sente davvero europeo e crede nel sogno di un Continente affratellato, come lo avevano pensato i padri fondatori, e pretende istituzioni all'altezza del compito, che sappiano interpretare i bisogni dei cittadini europei, che non si arrocchino a Bruxelles o a Strasburgo per perpetrare il loro potere. il loro potere. Chi fa queste critiche si aspetta di non essere rimbrottato da un qualunque commissario europeo che pretende di insegnarci a votare (una cosa grave). Chi crede nel sogno europeo e vuole più Europa non vuole avere a che fare solo con burocrati, ma vuole istituzioni democratiche, efficienti e attente, in cui la volontà popolare sia tenuta in massima considerazione. *(Applausi Signor Presidente del Consiglio, noi siamo una forza patriottica, responsabile e costruttiva che come tale si è comportata

che lei e anche i colleghi della maggioranza avete utilizzato finora in questo dibattito. Ciò a fronte delle dichiarazioni trionfalistiche, direi, purtroppo demagogiche e infondate, che lei fece subito dopo la riunione del Consiglio europeo, come se avesse vinto la Terza guerra mondiale. Sono passati quattro mesi e allora partiamo in modo concreto e, spero, che lei ci dica come è cambiato il paradigma europeo e italiano in questi quattro mesi. Come?

tra i punti approvati al Consiglio europeo rientravano maggiori sforzi per la nuova rotta mediterranea, più rimpatri volontari e accordi con Paesi di partenza e transito. Quali accordi sono stati realizzati in questi quattro mesi? quattro mesi? Sono aumentati i rimpatri e quanto? Ci dia dei dati su questi aspetti. L'Italia ha fatto nuovi accordi? L'Italia ha aumentato i rimpatri? proposito delle piattaforme di sbarco regionali e dei centri sorvegliati negli Stati membri, ancorché su base volontaria, ci spieghi in questi quattro mesi chi ha realizzato, tra i Paesi europei piattaforme di sbarco regionali e centri sorvegliati negli Stati membri. Ci spieghi se l'Italia lo ha fatto; fatto; altrimenti come si presenta in sede europea, dopo quattro mesi, se l'Italia per prima non fa nuovi accordi per il rimpatrio, se l'Italia per prima non aumenta i rimpatri, se l'Italia per prima non realizza piattaforme di sbarco regionali e centri sorvegliati? Come fa a rimproverare gli altri di non aver cambiato passo se noi non cambiamo passo? Per quanto riguarda i fondi, noi le chiediamo davvero che vi siano fondi di rimpatrio a carico dell'Unione europea almeno pari a quanto l'Unione europea ha dato alla Turchia per bloccare il fronte dell'est. Il senatore Stefano, che poco prima nominava alcuni Paesi dell'Europa centro-orientale che hanno tutelato la frontiera orientale d'Europa, come dimostrano numeri e fatti, si impegnano altrettanto nella frontiera mediterranea, forse dovrebbe nominare, invece, e declamare - lo dico anche al collega dei 5 Stelle - il Paese che ha sabotato - questo sì davvero il Mediterraneo e che agisce ogni giorno per far saltare ogni accordo sulla Libia; il Paese che sfrutta non le ex colonie ma le colonie africane,

Ha nominato i nuovi vertici dei servizi segreti o sono ancora transitori? Come affronta questa Conferenza senza prima risolvere i nostri problemi nei rapporti con la Libia e sulla sicurezza? Bene, le diamo Bene, le diamo un suggerimento: lei è stato nel Corno d'Africa e credo che sia importante per l'Italia attivare subito il piano europeo per gli investimenti esterni, che è veramente necessario ma ancora non è stato applicato. Soprattutto le consiglio di chiedere all'Unione europea che sia realizzato l'accordo di *partnership* economica con i Paesi del Corno d'Africa, così da consentire l'accesso al mercato, il commercio, le regole d'origine. Quello che necessita al Corno d'Africa - tra l'altro principale fonte di immigrazione - è sfruttare appieno il processo di pace. L'Italia può agire, può agire l'Unione europea e ci aspettiamo che lo faccia.

ma dal punto di vista degli interessi italiani. In questo momento il primo interesse italiano è che nell'accordo di recesso - e sottolineo accordo di recesso - e non nel successivo accordo commerciale che chissà quando vedrà la luce, vedrà la luce, sia posta in modo chiaro la questione di principio del riconoscimento delle indicazioni geografiche senza le quali si pregiudica il mercato del Regno Unito, uno dei primi al mondo, al nostro *made in Italy*. Il ministro Centinaio dovrebbe saperlo: allo stato non è così, allo stato nell'accordo di recesso siglato o comunque discusso fino a questo momento, non ci sono i riconoscimenti necessari delle indicazioni geografiche. Noi chiediamo che il Governo dica in maniera esplicita - in questa fase non dopo, quando sarà impossibile recuperare - nell'accordo commerciale che noi non firmeremo alcun accordo di recesso, non daremo il nostro consenso se in questo documento non vi sarà il riconoscimento dell'indicazione geografica, altrimenti avrete tradito gli interessi nazionali italiani per subordinarli ad una declamazione di principio ideologico. Infine, vengo alla Russia.

l'immediata cessazione delle sanzioni economiche imposte alla Russia, il prolungamento delle quali avrebbe il solo effetto di ampliare le già pesanti ricadute negative sulle nostre imprese»; nel Consiglio europeo del

purtroppo non corrispondono ai fatti. Noi crediamo che vi sia un Governo del cambiamento - del cambiamento per davvero - se alle parole corrispondono i fatti e se agli impegni corrispondono le azioni. Altrimenti, quando si cambiano

il Consiglio europeo dei prossimi giorni affronterà questioni che si trascinano da anni, *in primis* - lo sappiamo e lo abbiamo sentito anche in questa Aula - si discuterà dell'immigrazione. Abbiamo avuto ieri la conferma di come la Francia risolva il problema dei cosiddetti movimenti secondari da fare all'interno dell'Unione: ha caricato due migranti e li ha tranquillamente riportati in Italia, come se fossero italiani, come se un Regolamento assolutamente sbagliato, quello di Dublino, potesse cambiare il modo di vivere di un'Unione europea, il cui meccanismo di coesione scricchiola purtroppo sempre di più. il Regolamento deve essere modificato perché l'Europa deve condividere con l'Italia non sono le regole di bilancio, ma anche il peso di questo straordinario fenomeno epocale. è questo il primo mandato che lei dovrà affrontare nei prossimi giorni a Bruxelles. Il respingimento di ieri a Claviere, in Val di Susa, ci ricorda che abbiamo un argomento molto forte per fare pressione sull'Europa e, al contempo, un problema enorme da risolvere in Italia. un altro tema per il Governo che riguarda appunto la Val di Susa, dove - vorrei ricordarlo incidentalmente ai rappresentanti dell'Esecutivo - c'è un'opera importantissima strategica per l'Italia, per la quale si sono già spesi ingenti risorse, che riguarda i rapporti con la Francia e i movimenti di merci da e per l'Europa, ferma incomprensibilmente per i veti di una componente di questo Governo. Alcuni Paesi europei vogliono regolamentare in modo più restrittivo i movimenti secondari dei migranti ma, Presidente Conte, è l'Italia che si trova sul proprio territorio 630.000 migranti, che non hanno titolo alcuno per restare e che, pertanto, sono da considerarsi a tutti gli effetti clandestini. Si tratta di un numero destinato ad aumentare, perché sono ancora più di un centinaio di migliaia le domande di asilo da esaminare e sappiamo già che la più parte di queste - il 90 per cento almeno - non verranno accolte. Grazie anche a quella parte di programma del centrodestra che prevedeva l'abolizione della protezione umanitaria, ora opportunamente inserita nel cosiddetto decreto sicurezza, forse potremo avere qualche elemento in più di valutazione positiva. Un istituto, quello della protezione umanitaria, che però non esiste nel resto d'Europa e, quindi, non viene riconosciuto ai fini dei movimenti secondari di coloro che non sono considerati bisognosi di asilo: un autentico esercito di persone giunte in Italia, in quanto confine meridionale dell'Europa. Quindi, se l'Europa esiste, non può non farsi carico di un problema che è dentro i propri confini, dopo che ha mancato di vigilare. I confini vanno rispettati. A proposito, ci domandiamo, presidente Conte, se i confini esistano ancora. Se la risposta e sì, questi confini vanno garantiti e difesi. Prima di approvare qualsiasi disposizione che imponga all'Italia il riaccoglimento dei migranti da Francia, Austria, Germania o altri Paesi del Nord Europa, è necessario risolvere questo, che è un enorme problema sociale.

quale degli 8.000 sindaci in Italia non vorrebbe avere 1.050 euro per ciascuno dei propri abitanti, per i propri anziani, per i disabili, per i ragazzi?

che abbiano contributi e redditi molto bassi (anche perché spesso accettano parte di salario in nero) fa sì che sorpassino irresponsabilmente gli italiani in tutte le graduatorie. sono tra i primi nelle case popolari e nei servizi sociali e godono di esenzioni cui gli italiani più poveri non possono accedere. È giustizia sociale questa? È questo che noi chiediamo, signor Presidente.

Infatti, se il sistema di *welfare* corrispondesse alle tasse versate, ad esempio per il caso Lodi non avremmo dovuto dire, come ha fatto qualcuno, che paghino tutti. Bisognava dire: «che non paghi nessuno, né gli italiani, né gli stranieri se sono regolari e vivono in modo permanente in Italia e hanno famiglia». *(Applausi dal ora che abbiamo visto la manovra per il 2019, lo diciamo noi. Gli asili nido non ci sono e le scuole materne scaricano parte degli oneri sulle famiglie. Questi sono i primi interventi che avrebbe dovuto mettere in campo un Governo serio e sbatterli in faccia all'Europa. Un Esecutivo che avesse voluto avere il plauso dell'Europa, ma prima ancora degli italiani avrebbe dovuto dire: stiamo lavorando per ridare soldi ai Comuni italiani affinché le famiglie non debbano pagare nulla fino alla scuola dell'obbligo. Invece, viene ora introdotto il reddito di cittadinanza, una misura che si muove nell'alveo di un assistenzialismo che noi giudichiamo pericoloso per un Paese che, al contrario, avrebbe necessità di lavoro, aiuto alle imprese e alla produzione nazionale. Prima i nostri Comuni, prima i servizi resi alle nostre comunità, prima gli italiani. Anche il Sud ha una montagna di risorse: più di 50 miliardi che arrivano dall'Europa sono fermi perché i progetti che vengono presentati sono per lo più basati corrente e, quindi, non vengono accettati dall'Unione europea. Ecco, presidente Conte, le questioni che deve portare in Europa sono quelle relative alla condivisione di un problema gigantesco, quello della sistemazione di 630.000 persone, di cui l'Europa dovrà pure farsi carico. È quindi necessario un piano di rimpatri serio, forte e davvero condiviso da parte dell'Europa su un piano economico e organizzativo, accompagnato da una presenza importante dell'Unione europea in Africa, nei Paesi da dove viene la maggior parte dei migranti partiti da quel continente e giunti in Italia. Lo diciamo bene nella nostra proposta di risoluzione: la Cina ha investito sinora 125 miliardi di euro in Africa; altri 60 miliardi sono previsti nei prossimi tre anni attraverso linee di credito, aiuti e prestiti a tasso zero, fondi per lo sviluppo, e finanziamenti alle importazioni in Africa. L'Europa che si affaccia sul Mediterraneo non può aspettare, Presidente, di essere superata da altre economie quando l'Africa è a portata di mano e quando l'aiuto di quel continente può costare meno dei maggiori oneri sinora sostenuti per far fronte all'arrivo e all'accoglienza dei migranti. L'Africa può essere una gigantesca opportunità, ma vanno fecondati i rapporti economici, non la tratta degli esseri umani. Se pensiamo che lo scorso anno sono stati appostati, solo nel bilancio italiano, quasi 5 miliardi di euro, possiamo immaginare come sarebbero meglio utilizzate queste risorse economiche se messe assieme a quelle degli altri Paesi membri dell'Europa. Insomma, presidente Conte, un'altra chiave per risolvere il problema dell'Africa e della gente che scappa, molto spesso in cerca di migliori condizioni di vita, e mettere in piedi un serio piano di investimenti per l'Africa.

e di invitare i *leader* europei alla Conferenza di Palermo con uno spirito costruttivo e collaborativo, quello che Forza Italia ha messo in campo con la propria proposta di risoluzione, dettata da forte senso di responsabilità e da amore per la propria Patria.

Signor Presidente, i temi all'ordine del giorno del Consiglio europeo, dalle migrazioni alla sicurezza interna, alle relazioni esterne, alla Brexit, sino alle problematiche relative all'unione economica e monetaria, restituiranno ai nostri cittadini l'idea di quale Europa stiamo difendendo. Lo scenario internazionale ed economico nel quale si svolge questo Consiglio è sicuramente condizionato da nuove incertezze, con il diffondersi di politiche protezionistiche, a partire dagli Stati Uniti, con una ripresa economica che stenta ad affermarsi. Tuttavia, in tale quadro, l'Europa resta il mercato unico più grande del mondo, la principale potenza commerciale su scala globale, il primo donatore di aiuti umanitari allo sviluppo. L'Europa è il più vasto territorio guidato da democrazie. Per questo, crediamo che l'Unione europea non possa rinunciare a giocare un ruolo centrale nel mondo e in un contesto di geopolitica in divenire. Che l'Europa, dunque, torni a fare l'Europa nel quadro internazionale, ma anche nel processo di integrazione interna. In tale orizzonte, negli ultimi anni l'Italia si è posta in prima fila nella battaglia per la democratizzazione della *governance* e per la modifica sostanziale delle politiche di austerità, riuscendo a ottenere una significativa flessibilità, non solo a vantaggio del Paese Italia ma di tutti i Paesi membri, a sostegno degli investimenti, anche per invertire quel ciclo recessivo dell'economia di cui abbiamo potuto appena apprezzare gli effetti. Al contrario, la stessa vostra manovra economica sembra costituire una sfida alle istituzioni europee, un tentativo di bocciatura dei conti del nostro Paese che rischia di indebolire la stessa credibilità del Paese Italia. Nella stessa direzione vanno le conclusioni del Consiglio europeo di giugno, che hanno indebolito e vanificato nel loro complesso ciò che era stato portato avanti per rendere obbligatori i ricollocamenti dei migranti. Allo stesso modo non avete sostenuto la revisione del Regolamento di Dublino. Siete stati accanto ai Paesi di Visegrád contro gli interessi del nostro Paese nel recente vertice informale di Salisburgo, contro la proposta del potenziamento della guardia di frontiera per salvare l'accordo di Schengen, rafforzando Frontex e il diritto di asilo europeo. Non potete invocare più Europa, ma lavorare per meno Europa. Qual è dunque l'orizzonte verso il quale si state conducendo? Noi vogliamo un'Europa dei diritti, che sappia proteggere, che garantisca maggior sicurezza interna ed esterna, ma anche protezione e sicurezza sociale, prevedendo - e su questo siamo d'accordo - anche strumenti europei di lotta alle disuguaglianze e alle disparità territoriali, come previsto nel pilastro sociale europeo. un progetto politico per l'Europa che condizioni la dimensione economica; un'Europa che, dopo sessant'anni di pace e sviluppo, sappia stare vicino a quelle paure che caratterizzano anche la generazione di mio figlio. Spostiamo verso la dimensione europea il confine di tali istanze di sviluppo sostenibile, attento al cambiamento climatico, alla sicurezza interna ed esterna, anche a tutela di quella ricchezza culturale e identitaria dell'Europa a salvaguardia delle nostre democrazie liberali e contro le nuove forze della disgregazione sovraniste e nazionaliste. Voi state creando le condizioni per il divorzio dall'Europa. L'Europa non può essere il capro espiatorio dei vostri fallimenti. Ci state portando fuori rotta, assumetevene la responsabilità. Da parte nostra nessun vento contrario ci farà cambiare l'orizzonte verso quell'Europa politica, dei popoli e della democrazia.

sicuramente non l'abbiamo noi di Forza Italia. Io ho una carriera di giornalista alle spalle e da giornalista ho sempre criticato l'Unione europea, quando ancora andava di moda dirsi europeisti e quando, tra i popoli europei, quello italiano era il più europeista di tutti. Ad aprirmi gli occhi fu il presidente emerito Francesco Cossiga, il quale un giorno (ancora eravamo lontani dall'inizio della crisi economica) mi disse che se le istituzioni europee fossero state prese così come erano e trapiantate nell'assetto costituzionale di uno qualsiasi degli Stati membri, i cittadini di quello Stato sarebbero scesi in piazza per protestare e, se le proteste non avessero ottenuto risultati, sarebbero saliti in montagna. C'è un problema evidente di legittimità democratica delle istituzioni europee. È un problema di mancanza di identità, natura e visione politica e non è un caso, ma una scelta. Jean Monnet, che dell'Europa unita fu il grande e illuminato architetto, negli anni Cinquanta annotò sui suoi diari che l'Europa doveva nascere all'insaputa dei popoli. È evidente che qualcosa che nasce all'insaputa dei popoli non ha né può avere sostanza politica: funziona finché le cose vanno bene, ma ai primi venti di crisi mostra la corda, la propria debolezza. Ci siamo, ci siamo ormai da parecchi anni. la cura a questa malattia non è l'invettiva, non è la "sbrasata", non è l'esibizione muscolare. La storia recente ci ha insegnato che i Governi che hanno cercato di percorrere questa strada non hanno fatto l'interesse nazionale. La cura a questa malattia si chiama «politica» ed è quella politica che voi giustamente imputate all'Europa come grande assente, che è anche assente dai ranghi del vostro Governo. Purtroppo siete simili ai vostri avversari: non riuscite ad avere un'identità, una cultura, radici politiche e una visione di sviluppo del Paese e questo indebolisce l'interesse nazionale. State commettendo il più classico degli errori, quello che nei manuali manuali di strategia militare viene indicato come il primo degli errori da non commettere: state combattendo una guerra su due fronti. L'Italia ha due problemi sostanziali in quest'epoca: l'immigrazione e l'economia, intesa come mancanza di sviluppo, quindi mancanza di creazione di posti di lavoro. La soluzione di entrambi questi problemi dipende dalla condivisione dell'Unione europea e dei *partner* europei, voi avete dichiarato guerra su entrambi i fronti. Temo che questo metta l'Italia nelle condizioni dell'asino di Buridano: c'è il rischio serio che non riusciate a raggiungere alcun risultato, né sul fronte dell'immigrazione, né sul fronte dei conti pubblici e dell'eventuale sviluppo del Paese. La vostra manovra è emblematica di questo vizio d'origine che vi portate dietro: manca di visione politica. Il problema non è il 2,4 percento Va bene, ha dei costi; questi costi li stiamo già pagando e probabilmente continueremo a pagarli in termini di aumento del costo del denaro e questo ricadrà sulle nostre piccole e medie aziende, ma si può anche accettare di sostenere quei costi, in ragione di una manovra che promuova lo sviluppo economico. Però non è questo il caso: la vostra è una manovra puramente elettorale, un *patchwork* di misure che nulla hanno a che vedere con l'interesse nazionale. C'è un condono, chiamato pace fiscale. Vi ostinate a chiamare *flat tax* quella che non è una *flat tax*, ma è semplicemente un allargamento del regime forfettario per le partite IVA. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Non è una *flat tax*: le aliquote sono tre, dunque smettetela di chiamarla *flat tax*, perché non ha niente a che vedere con quanto era scritto nel programma del centrodestra. Gli investimenti sono per 3 miliardi: nessuno può ragionevolmente pensare che con 3 miliardi si rimetta in moto l'economia e nessuno può ragionevolmente pensare che l'economia si rimetta in moto con un prelievo forzoso nelle tasche dei pensionati, un esproprio proletario di quelle pensioni che voi stessi giustamente avete detto - fino a ieri e fino a prima di assumere responsabilità di Governo

come purtroppo ormai è noto, si è concluso con un fallimento. Vi siete sentiti in dovere di bluffare, accampando risultati che, con tutta evidenza, non avete raggiunto. Nulla è cambiato da allora; anche questo dovrebbe servirvi da lezione. È vero che,

Il Regolamento di Dublino è ancora lì, i movimenti secondari non sono ancora condizionati agli accordi di riammissione, la frontiera sud dell'Europa è ancora solo la frontiera sud dell'Italia, l'Europa intesa come comunità non esiste e non si fa carico dei problemi. E allora smettetela di urlare, smettetela di cercare nemici, smettetela di indicare capri espiatori e colpevoli: indicate soluzioni, fate politica. noi di Forza Italia non da oggi, ma da sempre abbiamo nel cuore categorie come Nazione, interesse nazionale, Stato, Patria; non ci siamo improvvisati su questo fronte.

come bussola l'interesse nazionale e cercare di perseguire questo obiettivo con realismo, perché il realismo è l'unico metodo della buona politica. Non è questo il caso, purtroppo; non è questo il caso. Voi uscite dalla realtà, vivete in una realtà virtuale, condizionata dai *social*; vivete in un eterno presente, non avete alcuna prospettiva di futuro e, facendo così, ledete l'interesse nazionale. La supplica, allora, è: per carità di Patria, uscite da questo meccanismo e abbandonate l'ossessione del consenso. Ne avete tanto di consenso, tantissimo; usatelo e mettetelo a frutto, fate delle scelte nell'interesse del Paese! Il consenso non è un fine, è un mezzo per risolvere problemi concreti. Uscite dall'ossessione del consenso e fate politica, perché questa è l'unica maniera per contrapporsi in modo credibile a un'Unione europea che ha logiche ragionieristiche, che poi sono le stesse vostre logiche, le logiche di questa manovra economica. Uscite dall'ossessione del consenso, fate politica. Questo vuol dire solo una parola: assumetevi le vostre responsabilità.

in tanti anni - troppi - i Presidenti del Consiglio svolgevano la loro relazione, si alzavano e se ne andavano. Ringrazio lei e il suo Governo per l'attenzione che presta e il rispetto nei confronti del Parlamento. Perché la sua attenzione rende meno rituale questo appuntamento e diventa sfidante anche per noi fornirle le migliori osservazioni su un ordine del giorno ampio e articolato, che lei ha perfettamente illustrato prima, verso una reale, sostenibile e umanitaria strategia europea sull'ondata migratoria che preme al confine mediterraneo. La frontiera europea necessita di protezione europea, condivisa e solidale, piaccia o non piaccia a Paesi come la Francia dopo il blocco delle sue frontiere di qualche mese fa - lo ricordiamo tutti - oggi viene scoperta persino in flagranza di riprovevoli astuzie. E io mi auguro che il suo Governo renda giustizia a questo Paese chiedendo alla Francia di rispondere di queste scorrettezze. Comportamenti come questi, infatti, rendono di tutta evidenza la necessità di rivedere e ridiscutere regole dei mandati e delle operazioni di Frontex e le superate previsioni di Dublino, per sviluppare efficaci politiche di partenariato che concentrino, a nostro modo di vedere, tutte le risorse possibili dell'Unione proprio in quell'area del Mediterraneo fino a quando non sarà superata l'emergenza umanitaria, che troppe volte si trasforma in tragedia umanitaria. da una lettura attenta di quel Regolamento, che è in via di approvazione proprio in questi giorni, si nota che esso prevede risorse sparse nell'intero globo, dedicate persino ai rapporti tra l'Unione europea e aree come aree come quella dei Caraibi o dei territori d'Oltremare - tanto per restare in tema francese - che tutti sappiamo essere ciò che resta della loro *grandeur* colonialista, già puntualmente ricordata dal collega Urso. Ci permettiamo di far notare l'anacronismo di 1,5 miliardi di euro allocati in quell'area, cioè dalle parti di Guadalupe, quando al nostro Paese, per fronteggiare l'emergenza migratoria, l'Europa ha assegnato meno di 100 milioni di euro,

Di recente, il commissario Oettinger ci ha illustrato il quadro programmatico finanziario, dovendo ammettere che il dopo Brexit, del quale lei ha parlato, necessita di ulteriori risorse da parte dei Paesi e degli Stati membri, da parte di tutti, anche per pagare una burocrazia, quella europea, che pesa per 9 miliardi di euro, che non sono proprio bruscolini. Ma noi le chiediamo invece di difendere la PAC e non di difendere i 9 miliardi della burocrazia europea. Oppure, per tornare alla grande emergenza immigrazione, potremmo proporre l'impiego di quelle risorse, così competenti e qualificate, impegnate a misurare zucchine o ad obbligarti a svendere le nostre sofferenze finanziarie come le nostre aziende, per aiutare invece le sfortunate popolazioni dell'altra dell'altra sponda del Mediterraneo o dell'Africa subsahariana o di Paesi come la Nigeria che, nonostante le grandi ricchezze, esporta capitale umano per le più violente organizzazioni criminali. È rinviabile ancora, come ha ricordato lei prima, un grande piano di assistenza e di aiuti per quei Paesi e per impedire che l'Europa venga ulteriormente destabilizzata? Noi crediamo che non si possa più attendere, e che, invece che zucchine, invece che i Caraibi, oggi tutto vada concentrato in quel Mediterraneo che è frontiera d'Europa *(Applausi dai Gruppi* *L-SP-PSd'Az e M5S)*, e in quella frontiera ci siamo soprattutto noi ad aver pagato in questi anni un prezzo altissimo. Ma mi sia consentito di dedicare alcune riflessioni sul punto che farete in preparazione del prossimo vertice di dicembre, uno degli ultimi, signor Presidente, di questa Europa che sta per finire, alla vigilia delle elezioni del prossimo Parlamento Europeo. Parlerete di assetto istituzionale e di *governance*, speriamo di *politeia*, come auspica il ministro Savona, e noi con lui! Vede, noi facciamo i conti con un assetto regolatorio dominato dagli *input* compulsati dalle crisi prodotte dalle speculazioni finanziarie, ma che dovrebbe riprendere il filo dell'analisi giuridica - e so di parlare a un esperto - per non tradire o, peggio, vedere soccombere la costituzionalità stessa del funzionamento dell'Unione europea. In questo contesto giuridico, non risolto da Nizza e men che meno da Lisbona, ci si è illusi che l'adesione alla moneta unica fosse capace di garantire vantaggi per tutti: dagli Stati ai cittadini, dalla riduzione dei tassi di interesse ai vantaggi del mercato interno, alla stabilità dei prezzi. Che la materia fosse ostile a una rigorosa analisi giuridica si era già verificato alla prima rilevante controversia sottoposta alla Corte di giustizia. Nella sentenza sul Patto di stabilità del 2004, infatti, la Corte è in grande difficoltà nell'inquadrare secondo schemi giuridici una questione eminentemente politica, quale la procedura per disavanzo eccessivo di due importanti Stati membri come Francia e Germania. Ricordo solo che la Francia, incorsa poi successivamente nella reale procedure di infrazione per eccesso di *deficit*, ci è rimasta per nove lunghi anni, uscendone solo nel maggio di quest'anno. È storia recentissima, è cronaca: la cronaca di un'Europa strabica, perché questo dimostra che le regole si interpretano o si applicano a seconda delle simpatie politiche e che non ci sono - ahimè

O piuttosto batterci per ritrovare una visuale corretta, ampia, che riporti l'Europa a onorare i princìpi per i quali è nata: sviluppo, crescita, coesione, inclusione e giustizia sociale, per rafforzare le democrazie e la pace, quel bene preziosissimo che l'Europa finora ci ha garantito? Il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, signor Presidente, intende sostenere, insieme agli alleati, le scelte di Governo che vanno e andranno proprio nella direzione della crescita, in Italia come in Europa. Ma a lei, signor Presidente del Consiglio, affidiamo il compito più arduo: convincere altri Paesi a stringersi in una rinnovata alleanza per il salvataggio estremo dell'Europa, resa moribonda da medicine sbagliate, calcoli e regole sterili che hanno aumentato divari e disuguaglianze, fragilità e paura del domani. Ma l'Italia è un Paese fondatore e dovrà essere rifondatore con nuove alleanze. Presidente Conte, mi permetta di affidarle, per concludere, una domanda da porre al presidente della Commissione Juncker, che sono certo incontrerà

che il reddito medio *pro capite* degli Stati membri sia di circa 30.000 euro (e il nostro sta esattamente nella media) mentre quello del suo Paese, il Lussemburgo, sia di 121.000 euro *pro capite* E quel *dumping* fiscale concesso al Lussemburgo, sempre dagli strabici, è solo l'ultimo di tanti strabismi. E allora, a questi signori, che auspicano la lezione dei mercati agli italiani che non votano come garba loro, servono urgentemente un paio di occhiali, per correggere tutto quello strabismo e anche per aiutarli a leggere bene la nostra manovra di bilancio, necessaria per rimediare i danni da essi prodotti alla nostra economia e a salvare questa Europa ammalata, distratta molte volte e troppe volte cinica.

la invidio molto, perché, dopo tutte le cose che ho sentito oggi in Aula, ho riempito quasi cinque o sei fogli. Spero che si ricordi tutto quello che le abbiamo detto e non vada soltanto con il suo punto di vista, altrimenti sarebbe alquanto inutile stare una giornata qua. Mia mamma diceva sempre: è inutile che stai otto ore a studiare, se poi, quando ti interrogano, prendi quattro. Non vorrei che le accadesse la stessa cosa, quando andrà al Consiglio europeo. Detto questo, Presidente, cerco di ancorare la discussione di oggi a quello che accade sul territorio.

alquanto preoccupati da quello che sta accadendo. I temi all'ordine del giorno sono l'immigrazione, la questione della Brexit e dell'Irlanda, le banche e la manovra economica; tutto questo, mi creda, incide sensibilmente sulla credibilità del nostro Paese, ma non riguardo al suo Governo, ci mancherebbe altro: credo che il Governo in carica vada sostenuto comunque; apportare le necessarie modifiche, portare le proprie opinioni e punti di vista, cercare di articolare decisioni del Governo in funzione delle provenienze di ciascuno di noi e del Gruppo di appartenenza, al quale è tenuto a dare voce, ovviamente. Nel caso di Forza Italia, abbiamo tenuto sempre in considerazione una serie di questioni, come l'immigrazione.

ma non abbiamo avuto riscontro positivo rispetto a questo. E ancora, le do una notizia: forse dall'alto dello scranno di Palazzo Chigi non ci se ne accorge, ma nei parcheggi

l'Italia si è fermata. Perché l'edilizia stenta ancora a partire? Perché gli investimenti dall'estero, ai quali eravamo abituati qualche anno fa, non arrivano più? O meglio, perché si sono fermati da lungo tempo e non ripartono? Quali sono le motivazioni? Faccio un ragionamento banale:

però, a limitare molto le dichiarazioni dei suoi Ministri, in particolare di coloro i quali hanno funzioni d'indirizzo importante, soprattutto sull'aspetto economico, perché, ogni volta che aprono bocca, qualche investitore scappa o se qualcuno potrebbe decidere di venire a guardare l'Italia con interesse, se ne guarda bene dal farlo. Cercate di avere una voce unica: metta una regola al Consiglio dei Ministri e sia solo lei a dare indicazioni, perché mi pare il più moderato del gruppo, che può dare una voce unitaria e sola.

e la prego di dire ai suoi Ministri che quando sono qui in Aula e quando il Parlamento parla di questioni legate al Governo, nel rapporto tra Governo e Parlamento, devono restare ed essere presenti come fa lei, secondo l'esempio che lei e non uscire dopo che hanno svolto il loro intervento, perché purtroppo se oggi il Presidente del Consiglio resta, molti altri se ne vanno. Qualcuno viene trascinato via, senza voler fare la parodia del ministro Tria, che ultimamente viene trascinato via ovunque o gli viene spento il microfono perché magari ha da dire qualcosa di più di quello che potrebbe dire. E a me spiace moltissimo, perché probabilmente potremmo avere un dibattito più franco e più costruttivo nell'interesse esclusivo della Nazione, di quelle imprese e di quei cittadini che ci guardano con preoccupazione. *(Applausi

il ricordo di quel 5 giugno, quando lei entrava in quest'Aula per chiedere la fiducia per il suo Governo. Noi di quel giorno ricordiamo tutto: ricordiamo il suo respiro emozionato, ricordiamo l'atmosfera elettrica di un momento che si vestiva di un'eccezionale novità, perché per la prima volta in Europa due forze politiche di massa si combinavano tra loro abbandonando il vecchio schema della contrapposizione ideologica, per dar vita a un contratto un contratto di ammodernamento. Due differenti culture decidevano di collaborare e da questa collaborazione nasceva una sfida italiana, una sfida alla criminalità cibernetica, di cui parlava lei, Presidente, alla criminalità internazionale, una sfida al *business* dell'immigrazione, una sfida alle ferite di una crisi deflattiva che una finanza sregolata ha reso infinita. Ecco, quando lei è venuto quel giorno, insieme alla nostra fiducia noi sapevamo che per lei sarebbero arrivate giornate difficili, perché le dichiarazioni di guerra le erano già state consegnate, se si ricorda signor Presidente. Si diceva: «Saranno i mercati ad insegnare agli italiani come votare». Detto fatto, perché così è stato e non le nascondo, signor Presidente, che la settimana scorsa in quest'Aula qualcuno di noi ha avuto modo di cadere in uno sfogo dicendo: «Se in questo Paese i Governi e le leggi le fanno le agenzie *rating*, allora noi ci alziamo e ce ne andiamo». Era uno sfogo, non si preoccupi Presidente. Era lo sfogo di chi combatte tutti i giorni in quest'Aula per la sovranità parlamentare, ma io le dico, signor Presidente, che lei può pure riferire ai signori del Consiglio europeo che qualunque siano le sollecitazioni che dovessero arrivare, qualunque siano le interferenze, qualunque siano le pressioni che dovessimo ricevere, non ci sarà uno solo di noi che si alzerà dallo scranno per lasciare il campo alla dittatura degli algoritmi. Perché noi siamo diversi. Noi vogliamo essere diversi perché noi pratichiamo una politica che in qualche modo è la capacità di immaginare il futuro, creando le condizioni perché questo si verifichi. Noi vogliamo che lei a Bruxelles proprio questo: la forza della ragione e delle idee deve prevalere sui numeri e sulle percentuali. I pochi minuti che mi restano a disposizione, non li userò per parlarle di numeri o di

dalla Guardia costiera, ma anche dai sindaci e dai volontari ai quali quest'Assemblea non può lesinare un ringraziamento per tutto quello che stanno facendo. *(Applausi che, come è stato detto stamattina, il principio dello Stato di primo approdo deve essere superato. Qualcuno si chiedeva che cosa abbiamo fatto da questo punto di vista: abbiamo fatto tanto, perché sotto il profilo della legislazione nazionale, abbiamo finalmente razionalizzato, abbiamo riordinato quella intricatissima giungla che era il settore delle richieste di protezione e lo abbiamo fatto assecondando lo spirito della Costituzione. Abbiamo dato una risposta giuridica, caro collega di Forza Italia, a quel finto perbenismo che si lavava la coscienza raccogliendo questi sventurati dal mare, il cui dovere etico di soccorso, però, si fermava nel momento in cui questi esseri venivano sbarcati in un porto italiano. Dopodiché, in terraferma, la vita, il destino, la sorte, il futuro di questi sfortunati smetteva di essere un affare della politica perché diventava un affare della 'ndrangheta, perché diventava un affare di

che a Palermo il Mediterraneo diventi e ritorni a essere il crocevia della pace europea e che l'Europa non si chiuda nei suoi ristretti confini, con la speranza di riuscire a frenare un fenomeno immigratorio, che purtroppo è ineluttabile. In Africa, entro il 2030, i giovani sotto i diciotto anni saranno 750 milioni, ecco perché ho sorriso amareggiato ascoltando il collega Renzi dire che l'emergenza migranti è finita, i numeri sono tornati normali e che il Governo sta facendo dei flussi migratori un falso problema. Signori, dopo aver saccheggiato il continente africano e concentrato tutte le ricchezze in Europa, questi 750 milioni di giovani migreranno verso il Nord, perché li spinge quella che è la forza più antica della terra: la forza della sopravvivenza! Il fenomeno migratorio è un fatto inevitabile e noi abbiamo il dovere di chiedere che il principio dello Stato di primo approdo venga superato, ma dobbiamo chiederlo tutti insieme insieme in quest'Aula, se vogliamo davvero smetterla di guardare al quotidiano, al contingente, se cerchiamo davvero di sforzarci di vedere in quale direzione stanno evolvendo i fatti, perché questa è la politica che ti consente di rimanere connesso alla realtà, alla società e alla storia. Se davvero esiste un'Europa

Due brevissime considerazioni, una sul vertice euro che la attende a dicembre e una sulla Brexit. Da questo punto di vista, il documento sulla Politeia del ministro Savona e la nostra risoluzione di oggi le suggeriscono valide soluzioni per una *governance* più efficace. È indubbio però che le ricette europee, che ci hanno somministrato attraverso le politiche dell'abolizione dei diritti sociali, dell'*austerity* e della povertà sono state un fallimento. se anni e anni di politiche restrittive non hanno impedito il lievitare del debito pubblico italiano, il quale è cresciuto con sostanziale continuità, continuità, che cosa può farci pensare che continuare in questa direzione sia una buona soluzione? Ponga questa domanda ai signori di Bruxelles e vedrà che otterrà solo silenzi e spallucce. Bruxelles, sì, Bruxelles: qualcuno le ha chiesto con quali alleanze l'Italia ha intenzione di salire al Consiglio europeo. europeo. Con quali alleanze? Chi chiede e chi parla oggi di alleanze dimostra di non avere chiaro l'attuale quadro politico europeo. Signori, l'Europa come la ricordavate voi non esiste più. L'Europa oggi è una comunità intrisa di livore e di egoismi. Gli Stati del gruppo di Visegrád, di cui ho sentito parlare stamattina, non hanno un'idea politica alternativa, sono uniti solo dal terrore di essere nuovamente invasi dall'est e pensano di poter frenare questo fenomeno costruendo quegli stessi muri che avevano costruito nel 1600. È saltato tutto, come si dice; sono saltati gli schemi, sono saltate le alleanze, sono saltate le intese e sapete perché? Perché questa Europa, così, non è utile è per questo che i britannici sono andati via, è proprio per questo: perché questa Europa della Grecia svenduta all'asta, del *dumping* fiscale di Olanda, Belgio e Lussemburgo, questa Europa del *surplus* *record* della bilancia commerciale tedesca, non interessa a nessuno. Non è utile per nessuno. Ecco che allora, piuttosto che parlare di alleanze - e mi accingo a concludere, signor Presidente - è necessario tessere, come ho sentito, un piano di rifondazione. Occorre, da parte di tutti noi, un discorso progettuale perché l'Europa torni più equa, più solidale, più vicina alla gente. Ed è in questa chiave costruttiva che

sessant'anni fa, nel 1957, noi siamo disposti nuovamente a sederci intorno ad un tavolo per disegnare la nuova architettura istituzionale europea. Dica, Presidente, che tutto ha avuto inizio in questa città e che in questa città possiamo ricominciare, perché in questa città è nato e morto Altiero Spinelli, che una volta disse: «La via da percorrere non è facile né sicura, ma deve essere percorsa e lo sarà». *(Applausi dai Dichiaro chiusa la discussione Comunico che sono state presentate le seguenti proposte di risoluzione:

signor Presidente del Consiglio, siamo contenti che lei abbia sottolineato l'importanza di un'Italia all'interno dell'Unione europea, ma alle sue parole devono seguire anche i fatti. Siamo d'accordo con il Presidente della Repubblica: abbassiamo i toni con l'Europa, perché le offese e le ingiurie creano solo imbarazzo. I territori che rappresenta in questo Gruppo credono nell'Europa, perché hanno provato sulla loro pelle il peso e il dolore dei muri e delle frontiere. Siamo europeisti perché crediamo si tratti dell'unica possibilità di contare qualcosa nel mondo globale e, soprattutto, siamo convinti che solo un'Europa unita ci garantirà, anche per il futuro, pace e benessere. Le offese non servono a nulla, come dimostra quanto accaduto in giugno, quando, con una strategia incomprensibile, l'Italia ha fatto un regalo ai Paesi di Visegrád con la ricollocazione facoltativa e non più obbligatoria dei richiedenti asilo. un clamoroso balzo all'indietro rispetto alle prerogative e alle necessità del Paese. Ricordiamoci sempre che la spinta verso l'Europa nasceva nella convinzione che, agganciando il Paese a questo treno, si sarebbero corrette storture, rese più moderne le istituzioni e l'economia, offerte maggiori opportunità ai cittadini. Certo, questa strada si è rivelata molto più tortuosa e difficile del previsto. Ma senza l'Europa, chissà se l'Italia si sarebbe mai liberata da alcuni suoi vizi storici: lo Stato-imprenditore con aziende che alimentavano assistenzialismo; le manovre finanziarie che ingrossavano il debito pubblico; i mercati chiusi, ai limiti del regime monopolistico, con discapito per i cittadini consumatori. Avete deciso di ricadere in uno di questi antichi vizi, il peggiore, quello del debito pubblico. E, intanto, si attacca l'Europa che fa notare tutto questo, proprio come quando davanti alla febbre ce la si prende con il termometro. La verità è che in questi pochi mesi l'Italia sta scivolando in una condizione di sempre maggiore isolamento. Presidente Conte, il nostro Gruppo ha sempre espresso apprezzamento per la sua persona. Dall'inizio lei aveva un compito difficile. Oggi ci chiediamo se rientra davvero nelle sue possibilità governare con responsabilità, senza assecondare pulsioni che guardano solo al tornaconto elettorale. Ma lei sta andando a un vertice internazionale in cui rappresenta tutto il Paese e, allora, auspichiamo che rappresenti anche quella parte della popolazione che chiede un altro approccio nei confronti dell'Europa e delle sue istituzioni e, soprattutto, un altro stile. Noi, da convinti europeisti, non possiamo che dirci preoccupati per quanto sta accadendo.

Nessuno trarrà benefici da queste chiusure, noi per primi, visto che siamo Paese di primo approdo e che abbiamo uno dei peggiori rapporti tra debito e PIL e proprio i vostri alleati sono stati i primi a rimproverarvi per lo scostamento del 2,4 per cento. Il voto di Libero e Uguali sarà un voto contrario alla vostra idea di sicurezza. Non sarà alzando muri e allargando le maglie della legittima difesa e negando visti umanitari che le cittadine e cittadini saranno più sicuri, ma investendo in servizi, trasporti, illuminazione stradale, stabilità e messa a norma degli edifici scolastici, interventi per le zone colpite dal sisma e da altre calamità, conversione ecologica, aiuti alle famiglie, incentivi all'assunzione, investimenti in *welfare* e in diritto allo studio. Un Paese sicuro è un Paese in cui lo Stato si preoccupa di tutti, in particolar modo degli ultimi, e ricuce il tessuto sociale. Voi lo state strappando sempre di più, giorno per giorno. E non saranno i figuranti sotto i balconi a portarvi in trionfo: le vostre false promesse stanno già mostrando la corda. Il voto di Liberi e Uguali sarà un voto contrario a ciò che siete e rappresentate: una squadra di incompetenti, che inventa *tunnel* dove non esistono; che a Genova immagina la ricostruzione di un ponte come luogo di incontro dove le persone possono vivere, giocare e mangiare, piuttosto che un ponte utile ai trasporti; che nega l'accesso alla mensa e ai libri alle bambine e ai bambini che studiano nel nostro Paese;

che colpisce invece di difendere; che attacca invece di curare; che guarda indietro invece che guardare avanti. Il voto di Liberi e Uguali sarà contrario a questo Governo e a favore di un Paese più giusto, più accogliente, più solidale e più umano, tutto quello che voi non siete e non rappresentate.

Nell'ultimo Consiglio europeo del 28 e 29 giugno scorso, molti giornali si sono soffermati sul *gossip* e su immagini di lei fotografato da solo e non particolarmente in sintonia con gli altri *Premier* europei. Ebbene, è stata un'immagine di gran lunga migliore di quella che eravamo abituati a vedere prima, con grandi sorrisi e pacche sulle spalle che poi nascondevano, di solito, grandi fregature. Erano i sorrisi che si è abituati a vedere sui volti dei giocatori esperti di *poker*, felici di aver trovato il pollo di turno da mettere in mezzo e fregare a fine serata. Si ricordi sempre dei *Premier* che l'hanno preceduta in quelle organizzazioni: quando le danno grandi pacche sulle spalle e sorrisi, la stanno fregando. Meglio essere antipatico ogni tanto, ma difendere gli interessi nazionali.

illustrare i diversi punti. Il primo, fondamentale, riguarda l'immigrazione. Il dibattito di oggi è stato importante, perché si sono chiarite delle posizioni. Purtroppo il presidente Grasso, il PD e anche il MoVimento 5 Stelle hanno parlato tutti con un'unica voce, che è molto diversa dall'impostazione di chi vuole difendere i confini esterni dell'Unione europea. Il Governo deve chiarirsi prima di andare al Consiglio europeo. Qual è

ha chiarito bene qual è la posizione del MoVimento 5 Stelle, che non è, però, la posizione di Fratelli d'Italia e non è la storica posizione della destra. Infatti, semplificando,

i cattivoni dell'Est - mi riferisco al gruppo di Visegrád e Orbán - non sono d'accordo sulla politica del farsi invadere, allora non sono nostri alleati. Noi invece siamo alleati di Orbán e del gruppo di Visegrád, perché sosteniamo che l'Italia e l'Europa debbano difendere i confini esterni dell'Unione europea. Ebbene, su questo, presidente Conte, lei deve avere le idee chiare. Non si può andare in Europa a dire contestualmente entrambe le cose. Facciamo entrare chi arriva, perché la pressione è ineluttabile, e mettiamoci d'accordo tra europei su come far entrare tutte queste masse di disperati, oppure controlliamo i confini esterni. Non possiamo dire entrambe le cose, perché poi, magari, è proprio questa ambiguità che fa sì che su determinati punti non ci capiamo. europeo è stato stabilito il controllo dei confini esterni dell'Unione europea; tuttavia, come abbiamo detto subito, ci sono dei problemi perché, per quanto riguarda il controllo delle frontiere del Mediterraneo centrale, vengono destinati solo i 500 milioni del fondo per l'Africa, mentre per la rotta balcanica, quindi quella che parte dalla Turchia, 3 miliardi. Abbiamo detto di cercare di raggiungere una proporzione più equa

poi, il grave problema che siamo inadempienti rispetto a quello che è stato detto al Consiglio europeo, dove è stato stabilito che chi entra illegalmente in uno degli Stati dell'Unione europea deve essere trattenuto in centri sorvegliati. Ce lo ha ricordato perfino la Commissione europea e noi continuiamo a non farlo. Visti gli interventi di oggi, anche del Gruppo MoVimento 5 Stelle, viene il sospetto che non lo facciamo perché non lo vogliamo fare. caso, ce lo vuole spiegare? Nel Consiglio europeo è stato stabilito che se una persona entra illegalmente può essere profugo, richiedente asilo, clandestino, un turista, qualunque cosa: deve essere trattenuto in un centro sorvegliato. La Germania lo ha già fatto; ha già attivato il primo centro in Baviera, dove chi entra illegalmente viene trattenuto per diciotto mesi. Perché l'Italia non lo fa? Perché ha la stessa visione di Macron, di Soros? Perché non lo fa? lo fa? Non possiamo contestualmente andare a fare i sovranisti e poi dire, con il MoVimento 5 Stelle, che dobbiamo fare entrare la gente e distribuirla in Europa.

presidente Conte, vorrei che lei, al prossimo Consiglio, ponesse sul tavolo il problema del franco francese africano. La Francia attualmente stampa la moneta per 14 Stati africani *ex* colonie. Questo non è un favore che la Francia fa a questi Paesi perché, in cambio, oltre a farsi dare gli interessi e fare opera di signoraggio, chiede il deposito del 50 per cento delle entrate provenienti dalle esportazioni. Quindi, per capirsi: uno Stato che vende alla Germania per un miliardo, deposita 500 milioni alla tesoreria francese. È facile fare i buonisti in questa condizione! Se vogliamo parlare di Africa, cominciamo a

dal 2004 al 2017 ci sono stati 10 attentati islamici in Europa, con 600 morti, 4.000 feriti. Parliamo di questo, quando parliamo di sicurezza dentro l'Unione europea, perché è un altro tema tabù all'interno dell'Unione europea: non si può parlare di islam, non si può parlare di terrorismo islamico. parliamo anche degli *hacker*, magari di quelli russi, ma concentriamoci su chi gli attentati e i morti li fa in Europa. Vedo che ho ancora un minuto sanzioni alla Russia, durante tutta la campagna elettorale abbiamo sentito le forze di maggioranza sostenere l'abolizione delle sanzioni alla Russia: il Governo lo ha ribadito, l'ha anche scritto nel programma di Governo. Fratelli d'Italia ne è felicissima, perché lo sostiene da sempre. Eppure, all'ultimo Consiglio, Conte, ha approvato le sanzioni alla Russia. Anche in questo caso, qual è la linea del Governo? Capiamoci subito, Fratelli d'Italia non è un movimento che guarda con simpatia alla Russia; noi siamo nazionalisti e non guardiamo con simpatia a nessuno,

Brexit, perché gli accordi Brexit non prevedono la tutela delle indicazioni geografiche italiane: se non vinciamo questa battaglia in fase di trattativa non riusciremo a farlo dopo. Invitiamo pertanto il Governo a valutare

signor Presidente del Consiglio, le dirò che le sue dichiarazioni non hanno sciolto il nodo di fondo che pesa sulle relazioni tra il Governo italiano e le istituzioni europee:

potrebbe anche decidersi di non partecipare più a riunioni di istituzioni europee fino alle prossime elezioni, perché solo la salvifica scadenza elettorale

congiura giudaico-massonica ordita da chissà chi e finalizzata a nullificare il libero esercizio democratico dei cittadini italiani, che - io concordo - è sovrano e va rispettato.

che il Regolamento di Dublino non sarà modificabile se non all'unanimità, perché nel Consiglio europeo c'è un blocco di Paesi, quelli sovranisti di Visegrad, che sono i vostri sodali politici, ma che non possono essere alleati dell'Italia se il Governo italiano vuole portare a casa alcune risposte positive sul tema dell'immigrazione. *(Applausi

al popolo africano; un piano che sia fatto innanzitutto di educazione, di imprenditoria giovanile, di dignità per le donne, di lotta alla violenza sessuale. Ma con quale alleanza facciamo a livello europeo questo piano? Con quelli che dicono che non gli importa niente dell'Africa e che gli interessa soltanto quanto succede in Ungheria o in Polonia? Polonia? L'asse geopolitico conta: nella storia è sempre stato importante avere un asse di riferimento in Europa. Anche sul tema della manovra economica, senatrice senatrice Bonfrisco - ma potrei rivolgermi a tanti altri amici - molti di noi in quest'Aula, di opposizione e di maggioranza, condividono il punto che il problema dell'Italia sia non il debito, ma la scarsa crescita. E lo voglio dire con forza. Ma, se questo è il problema; se siamo d'accordo persino sul fatto che non possiamo impiccarci ai decimali e agli algoritmi - noi siamo su questa posizione - e sul fatto che regole scritte una volta e per sempre non possono essere immodificabili, prescindendo dalle condizioni socio-economiche dei Paesi in cui quelle stesse regole devono essere attuate e se vogliamo avere e se vogliamo avere maggiori margini di manovra sul bilancio, bisogna fare quello che è stato fatto dai governi Gentiloni Silveri e Renzi, e cioè negoziare con la Commissione europea margini di flessibilità. Ma per fare cosa? Per fare non una manovra a debito per fare spesa corrente, bensì una manovra a debito per fare spese per infrastrutture. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Questo è il punto politico che dobbiamo avere il coraggio e la chiarezza di spiegare agli italiani. Si può fare debito? Certo che si può fare debito.

si rilancerà una politica per le piccole e medie imprese sulla sostenibilità ambientale, facendo poi tanta politica per l'educazione e per gli scambi giovanili. Questa è politica per la crescita. Ma di tutto ciò non c'è non c'è nulla o poco meno di nulla nel vostro Documento di economia e finanza. Quindi, caro presidente Conte, voi dovete fare chiarezza. Volete fare gli alleati di Orbán e di Kaczynski? A proposito, sarei molto curioso di sapere come voterà, quando in Consiglio si dovrà applicare l'articolo del Trattato a proposito dell'Ungheria e di Orbán, così come votato dal Parlamento europeo. Voi volete fare gli alleati politici di questi e poi volete portare avanti degli obiettivi sull'immigrazione, sull'Africa e sulla manovra economica che essi stessi non vi consentiranno, perché i primi avversari del debito sono proprio Chi può ascoltare una voce in termini di richiesta di flessibilità non sono gli amici del gruppo di Visegrád. Qui c'è la grande contraddizione politica del Governo italiano e delle due grandi forze che lo rappresentano.

Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, questo è un momento strategico importante per il nostro Paese e per l'Europa. Quello nel quale ci troviamo a operare è un contesto storico inedito, in cui il mondo globale, dove l'Unione europea riveste il ruolo di attore, sta mutando profondamente e l'Unione europea stessa sta attraversando un ciclo di forte fluidità politica e istituzionale. Questo è non un momento di stabilità, bensì un tempo di cambiamento e trasformazione. Ogni vertice europeo, formale o informale, negli ultimi anni si è trovato ad si è trovato ad affrontare problemi epocali e macro questioni culturali e socio-economiche, dimostrandosi tristemente inadatto a superare la dimensione emergenziale, a mettere in campo strategie vincenti sul medio e lungo periodo e a costruire il benessere di quei popoli europei che, nel segno di un'Europa pacificamente unita, hanno visto la speranza di un avvenire migliore di quanto sia stato il passato da cui proveniamo. Dal 2011 ad oggi, signor Presidente, ogni vertice europeo ha visto la partecipazione di un'Italia debole, sopraffatta dal complesso di essere l'ultima della classe e guidata da un'*élite* politica che di quel complesso ha fatto la bandiera della propria azione di Governo e della propria egemonia culturale. Oggi, tra i tanti cambiamenti avvenuti sullo scacchiere europeo, il più significativo è senza dubbio la presenza di un'Italia finalmente priva di complessi, finalmente consapevole della propria forza e decisamente orgogliosa delle nuove prospettive amministrative aperte dal voto popolare alle passate elezioni politiche nazionali. un'Italia senza più il cappello in mano, rappresentata con dignità e onore dal presidente Conte e dai suoi Ministri. È possibile che oggigiorno, grazie al dinamismo dell'Italia, sulla scena comunitaria, finora governata dall'asse franco-tedesco, vengano superate sia la dimensione emergenziale con cui certe problematiche sono state affrontate in passato; sia il regime di austerità economica imposto all'eurozona a partire dal 2011 con tutte le sue contraddizioni; sia quelle fratture in seno agli Stati europei, come la trattativa sulla Brexit, che rischiano di creare un'infausta rigidità nelle future relazioni internazionali. il prossimo vertice europeo, sul quale ci esprimiamo, avrà all'ordine del giorno queste enormi questioni. Il flusso migratorio verso l'Europa non può certo essere trascurato, soprattutto all'indomani di un periodo estivo durante il quale sono emersi due dati di fatto incontrovertibili.

In secondo luogo è stato dimostrato dal resto d'Europa che la solidarietà esiste solo a senso unico, e cioè dall'Italia verso gli altri Stati, e non dagli altri Stati verso l'Italia. venti immigrati della nave Diciotti sono stati presi dall'Albania, e non dalla Francia, la quale però non perde occasione per fare la morale. Non solo ci fa la morale, ma ci prende in giro, perché questa mattina Macron ha avuto il coraggio di dare la responsabilità agli agenti in quanto inesperti per l'invasione in territorio italiano. *(Applausi dai Gruppi*

L'unica è l'Italia, che finalmente mette in campo soluzioni durature, a medio e a lungo termine. Ma non possiamo essere lasciati soli, o meglio: chi decide di lasciarci soli deve sapere che su questa partita non ci vedrà disponibili a dialogare su altre problematiche. Un altro problema a cui sono state date scarse risposte è la lotta alla cybercriminalità, che aggredisce i mezzi di informazioni con lo scopo di tacitare o distorcere i messaggi delle istituzioni o di gruppi di opinione, turbando la libera circolazione delle idee, che è il cuore pulsante delle nostre democrazie. Sotto questo punto di vista non sono state prese che timide iniziative. Bisogna fare di più. Si profila all'orizzonte anche il vertice euro, nel quale verrà discussa l'integrazione economica europea e le sue prospettive future. Sarà un'occasione importantissima per smantellare il dogma dell'*austerity*. Il fallimento dell'*austerity* è sotto gli occhi di tutti, ma un punto di vista sul quale vorrei attirare l'attenzione dell'Assemblea è è che il regime di austerità ha portato alla disaffezione dei popoli non solo verso l'attuale assetto delle istituzioni europee, ma anche verso la stessa idea di Europa unita. Il germe dell'intolleranza tra Nazioni è tornato a serpeggiare, e ciò non a causa delle forze cosiddette populiste, che anzi sono le sole a credere ancora in un disegno europeo di popoli fratelli e liberi dalla dittatura finanziaria *(Applausi dai Gruppi*

c'è chi gioisce per gli attacchi alla democrazia; quella democrazia per cui molti hanno dato il sangue e che non sarà certo lo *spread* ad abolire. La Brexit, poi, ci riguarda da vicino. Sono stati trovati accordi di massima per quanto riguarda molti aspetti importanti, ma resta ancora insoluta la questione circa il confine tra Irlanda e Irlanda del Nord, nonché l'importante individuazione del tipo di partenariato economico-commerciale *post* Brexit. Sono aspetti molto controversi che fanno emergere lo spettro di un *nodeal* e delle turbolenti relazioni diplomatiche che ad esso seguirebbero. Sotto questo punto di vista, è nostro impegno imprescindibile salvaguardare la comunità italiana nel Regno Unito ed essere fermamente al fianco dell'Irlanda. In questo contesto, abbiamo una certezza alla quale non si intende venire meno, con buona pace di quanti fanno terrorismo mediatico al riguardo. Siamo fermamente all'interno dell'Alleanza atlantica che era, è e sarà l'imprescindibile schema bellico unitario dell'Europa. Concludendo, signor Presidente, sosteniamo fermamente l'Esecutivo nella richiesta di un rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione europea per evitare tragedie in mare; nella richiesta di una riforma oculata del Trattato di Dublino; nell'incoraggiare la cooperazione

Sosteniamo, altresì, la lotta alla cibercriminalità e alla criminalità organizzata e la volontà di promuovere tutte le iniziative necessarie per creare un gruppo di lavoro che studi l'attuale architettura europea e la politica economica europea, nell'ottica di rispondenza effettiva ai trattati, i quali affermano la crescita nella stabilità e l'aumento del benessere di tutti i cittadini europei, nessuno escluso. In ultimo, crediamo fermamente che questo Governo possa e debba attivarsi per fare della Banca centrale europea una vera banca sovrana, capace di svolgere il ruolo di prestatore di ultima istanza. Il fatto che si trovi materialmente a Francoforte la dice lunga sulla sua reale indipendenza. Disinneschiamo, infine, lo *spread*. Togliamo ai potentati economici, che nessuno ha mai votato, il potere di destabilizzare le democrazie e silenziare i popoli sovrani. Per questo motivo, il Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier- Partito Sardo d'Azione, voterà convintamente la risoluzione, nella consapevolezza di operare per dare nuovamente sovranità e dignità ai popoli europei oppressi e affamati.

il 5 ottobre scorso i commissari europei Dombrovskis e Moscovici hanno scritto una lettera al Ministro dell'economia italiano criticando duramente la Nota di aggiornamento del DEF, perché si discostava dalle raccomandazioni approvate dal Consiglio europeo per quanto riguarda il rientro dal *deficit*. Quella lettera è stata accolta da durissimi attacchi da parte di esponenti del Governo e della maggioranza

coloro che vogliono imporre la dittatura degli algoritmi". Chissà quale Consiglio europeo aveva approvato quelle raccomandazioni, anche perché erano state approvate all'unanimità e, dunque, anche con il voto dell'Italia.

E invece no, perché quel Consiglio europeo si è tenuto non nel passato ma il 28 giugno scorso e a rappresentare l'Italia e a votare quelle raccomandazioni c'era il qui presente presidente del Consiglio Giuseppe Conte. *(Applausi

non credo che a livello europeo questo dia credibilità al nostro Paese, specialmente poi se abbinato a ferocissimi attacchi contro i cattivoni del Consiglio europeo, per non parlare dei componenti della Commissione europea, che - a detta di esponenti del Governo

molti interventi senza prendere appunti si rischia di non ricordare molto, ha fatto un'osservazione davvero appropriata. Sono infatti passati tre mesi da quelle raccomandazioni e lei ha firmato una Nota di aggiornamento al DEF e una legge di bilancio che si scontrano frontalmente con quelle raccomandazioni.

qui lei ha ricevuto la raccomandazione - anzi, l'impegno - da parte della maggioranza di Governo - e, su alcuni punti, anche di altre forze politiche a lavorare su alcuni aspetti, come l'eliminazione delle sanzioni alla Russia, che fanno più danno a chi le pone che a chi le riceve

Purtroppo è bastato che trascorresse qualche giorno perché la vicenda della nave Diciotti ci facesse scoprire che non avevamo ottenuto assolutamente nulla, neppure dal punto di vista dell'immigrazione: le persone che erano a bordo di quella nave

Qui poi subentra la questione della manovra, della quale ha parlato e che si scontra con le raccomandazioni approvate dal Consiglio europeo, anche con il suo voto, il 28 giugno; ma questo ormai l'abbiamo visto, questa manovra non ci pone nella direzione giusta né nelle condizioni di imporci a quel pericoloso organismo che si chiama Consiglio europeo o alla Commissione europea. invece in una condizione d'isolamento, perché metterci frontalmente contro a quanto era stato chiesto all'Italia,

anche speculativi e politici, per non parlare di quelli giudiziari; ha però difeso l'Italia, cercando sempre il dialogo con gli altri Paesi. Non possiamo attaccare

immigrati, per il resto non abbiamo tante cose in comune. Possiamo avere tanta simpatia e alcune vedute in comune: se però non vogliono prendersi nessuno dei nostri immigrati, che noi invece vogliamo dare loro, non vedo il grande interesse in comune. comune. L'isolamento che invece abbiamo oggi era esattamente l'opposto di quello che Silvio Berlusconi ha sempre portato avanti con i suoi Governi, ottenendo cose notevoli, di cui adesso non faccio l'elenco, limitandomi a parlare solo dei successi ottenuti proprio per attutire quelle norme eccessivamente rigide e difendere gli interessi dell'Italia, il *made in Italy* e tante altre questioni.

direttiva Bolkestein dove non va applicata; quando si batterà per difendere i confini dall'immigrazione clandestina e anche dalle incursioni che vengono dalla Francia; quando difenderà gli interessi dell'Italia e la sicurezza dei cittadini;

un ottimo trattamento; ma allora impariamo, imparate qualcosa anche da Trump. Trump, da quando è stato eletto, ha fatto salire i valori della Borsa americana del 40 per cento e la disoccupazione è ai minimi. Da quando

è in aumento. Prenda esempio dall'unico punto di riferimento che - a quanto pare - questo Governo è riuscito in qualche modo ad avere, forse più che altro per via del nemico comune che è la Commissione europea, e cerchi di fare l'interesse dell'Italia. Signor Presidente, presidente Conte, membri del Governo, colleghe e colleghi, anche oggi ci troviamo qui a parlare d'Europa

l'Europa ha deciso di lasciare agli Stati membri tutta la sovranità su temi come l'immigrazione, dove invece serve una sovranità europea, e ha deciso invece di tenere per sé la sovranità economica e finanziaria, laddove invece all'interno degli Stati membri servono totale sovranità e autonomia. Esempi di come quella sovranità nazionale per affrontare temi di carattere europeo dimostra tutta la sua fragilità, e e quindi che poi il rapporto tra gli Stati membri si basa su egoismi, li abbiamo quasi quotidianamente: abbiamo visto quello che è successo ieri nel rapporto con la Francia; abbiamo visto la Gendarmeria francese portare sul nostro territorio gli immigrati; l'abbiamo visto a Bardonecchia; l'abbiamo visto molte volte nel Mediterraneo, quando Stati membri chiudono i propri porti pur avendo l'obbligo di andare a salvare vite umane. Su questo però la sovranità è sempre in capo ai popoli. E lo vedo ogni giorno sul mio territorio: se ne parla pochissimo, dalla frontiera del Friuli-Venezia Giulia entrano ogni giorno centinaia di persone. E non se ne parla perché non arrivano su una barca. Io, però, che ho studiato geografia al liceo credo di ricordare che intorno al mio confine si trovano tutti Paesi membri dell'Unione europea e mi chiedo allora come mai è sempre l'Italia a doversi fare carico di tali arrivi.

senatore Pittella ha fatto riferimento ad accordi che devono essere fatti con l'Europa per chiedere maggiore flessibilità, maggiori interventi e maggiori impegni finanziari. Io, però, mi chiedo come sono stati fatti tali accordi, perché l'Italia è il Paese che ha saputo uscire dalla crisi

presupposto sbagliato, di questo paradosso di mancanza di sovranità - da un lato - e di abbandono di sovranità - dall'altro - i cittadini si trovano ovviamente disorientati e non capiscono bene a che cosa serva questa Europa.

studi giuridici, ma credo che l'articolo 1 della Costituzione affermi che la sovranità appartiene al popolo ed è lì che ci sono i concetti di sovranismo e pupulismo che piacciono a questa maggioranza. Credo invece che il Governo, grazie all'ottimo lavoro del presidente Conte, stia facendo recuperare all'Italia quel ruolo importante che ha in Europa, come è stato ricordato dall'intervento del senatore Licheri. L'Italia è uno dei Paesi fondatori di quella che era la Comunità europea ed è sul concetto di comunità che dobbiamo insistere, sul concetto di aiuto tra popoli diversi, che hanno caratteristiche diverse, che vogliono essere sovrani su certe cose, ma che hanno bisogno gli uni degli altri per affrontare temi che singoli Paesi non riescono ad affrontare e hanno bisogno dei *partner* europei per affrontarli assieme non in una lotta dove vincono o perdono i sovranismi, ma in una

ma ai cittadini che vivono in quei territori e che hanno bisogno di avere chiarezze e certezze da un ente come quello europeo che, nel suo insieme, ha la possibilità di affrontare anche grandi problemi quale quello dell'immigrazione. Presidente Conte, noi votiamo a favore della risoluzione di maggioranza e la maggioranza sarà al suo fianco nel Consiglio europeo, perché credo che i temi che lei vuole portare in quel luogo sono quelli che giustamente dobbiamo affrontare in modo coeso.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

abbassare sensibilmente il volume delle conversazioni e lasciare libero il banco del Governo.

recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni

lo stesso Presidente della Repubblica, nonostante alcune modifiche apportate nella stesura finale del decreto‑legge, contestualmente alla firma del provvedimento ha fatto recapitare una lettera al Presidente del Consiglio, in cui chiede il rispetto degli obblighi costituzionali, in particolare dell'articolo 10

quanto sia fondamentale, nell'esame di questo decreto-legge, tener presente che c'è l'articolo 10 della Costituzione, che fino a oggi certamente non è stato abolito.

Lo dico con forza perché siamo pieni di dichiarazioni del Ministro dell'interno, il vice*premier* Salvini, che, con tutti i suoi strumenti di propaganda, continua a dire che si è ridotto sensibilmente il numero degli arrivi e effettivamente, il numero

devono essere chiare e non oggetto di mere intenzioni, perché politicamente si ritiene che bisogna intervenire con un decreto-legge.

l'omogeneità non è certamente rintracciabile: un coacervo di misure amministrative che intervengono su diversi temi, dall'immigrazione all'agenzia per i beni sequestrati, ai blocchi stradali, alle misure per le Forze dell'ordine. Aver, poi, utilizzato la parola «sicurezza»

colpevolezza, perché l'immigrazione, secondo questo decreto-legge, è semplicemente un problema di sicurezza pubblica.

e gli strumenti che uno Stato democratico deve mettere in atto. Il diritto d'asilo, che è garantito dal terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione, non viene adempiuto solo recependo il diritto europeo per quanto riguarda lo *status* di rifugiato e la protezione sussidiaria, ma soprattutto applicando concretamente una protezione umanitaria dello straniero; quindi, la sua abolizione di fatto viola la richiamata disposizione costituzionale. È evidente e anche nella sentenza della Cassazione del 2018 si dice con chiarezza che lo strumento della protezione umanitaria non è residuale, nel senso che dovrebbe essere elemento accessorio, ma è elemento che trae la sua forza e la sua provenienza direttamente dall'articolo 10 della nostra Costituzione. Al posto della protezione che cosa si fa? Si introducono

Ma guardate che il fatto di tipicizzare, quindi di incanalarli solo in alcune fattispecie, non esaurisce il richiamo dell'articolo 10 della Costituzione, che ci obbliga, non solo moralmente, ma anche dal punto di vista del fondamento del nostro patto repubblicano, a rispettare e ad avere il diritto d'asilo e la protezione umanitaria tra i valori fondanti della Repubblica, per non parlare di tutte

la revoca della cittadinanza a coloro che si siano macchiati di crimini e di reati molto pesanti. Si introduce una discriminazione, in violazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione, tra

Presidente, è una violazione acclarata e palese dell'articolo 3 della Costituzione. Ci sono cittadini italiani, che lo sono per nascita, per sangue, che si sono macchiati di delitti efferati e mantengono la cittadinanza, ovviamente, e

della Costituzione. Si introduce un trattenimento ai soli fini dell'identificazione per trenta giorni e, se non si è identificato, per altri centottanta giorni, con palese violazione di di vari articoli (2, 3, 10, 13 e 117) della nostra Costituzione, tra l'altro provvedendo a trattenimenti in luoghi non ben identificati, con tutto quello che significa dal punto di vista della libertà personale. Non si può avere avere una discriminazione così palese. Concludo, Presidente, ricordando che oggi è il 16 ottobre: dovremmo ricordarci tutti che è l'anniversario della deportazione degli ebrei dal ghetto di Roma. Noi, ancora ancora una volta, nella storia di questo Paese, stiamo compiendo atti palesemente discriminatori per razza, per nascita e per appartenenza;

Signor Presidente, anch'io, come la collega De Petris, sono rimasto molto colpito dalle audizioni che abbiamo svolto - ancora non sono terminate quelle programmate - in Commissione affari costituzionali. La ragione per cui sono rimasto molto colpito dai pareri che abbiamo ascoltato è che la quantità di elementi che all'interno di questo decreto-legge si pongono in aperto contrasto con articoli della nostra Costituzione, con sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenze e ordinanze della Corte di cassazione e con sentenze della Corte costituzionale sono veramente tanti. Noi intendiamo utilizzare il tempo che ci è concesso per l'illustrazione della nostra questione pregiudiziale per rivolgere un appello alla maggioranza, affinché riconsideri l'opportunità di procedere con l'iniziativa legislativa in esame. Alla luce di quello che abbiamo sentito,

da indurci a pensare che di questo provvedimento non rimarrà in piedi niente, non appena chi è adibito ad esercitare il controllo di legittimità costituzionale sugli atti del Parlamento lo esaminerà e prenderà una decisione sulla sua conformità alla Costituzione.

i problemi con misure efficaci e di non cedere alla tentazione della demagogia. Ci sono davvero aspetti che lasciano sconcertati: è stato ricordato il contrasto palese con l'articolo 10 della Costituzione del punto del provvedimento che prende il nome dal Ministro dell'interno e che prevede l'abolizione della protezione umanitaria. grossissimi dubbi le questioni del trattenimento per l'identificazione, dell'allungamento da novanta a centottanta giorni del periodo di permanenza nei centri per il rimpatrio, dell'esclusione dalla possibilità di registrarsi all'anagrafe per le persone che chiedono asilo, che significa l'esclusione di una categoria di persone dal godimento di diritti sociali fondamentali. Rilevanti perplessità sono suscitate anche dalla norma sulla revoca della cittadinanza. Durante le audizioni, uno dei costituzionalisti che abbiamo ascoltato ha citato una bellissima affermazione, fatta in sede di Assemblea costituente, da un grande padre costituente veneto, Umberto Merlin, che disse che lo Stato, contro i cittadini indegni, ha sempre altri mezzi di difesa più degni della revoca della cittadinanza, che non è mai tollerabile. Grandi perplessità sono sollevate anche dal fatto che la clausola di invarianza finanziaria, scritta nel provvedimento, è palesemente incompatibile con le norme contenute nel provvedimento stesso, che sono destinate a produrre aggravi burocratici, amministrativi e anche finanziari, oltre ai profili profili di illegittimità che ho appena ricordato. E poi guardate, il rischio maggiore, che ci fa propendere per la richiesta di non passare all'esame del provvedimento, è che si sia di fronte ad un atto che fa esattamente il contrario di quello che si propone, che ottiene effetti opposti a quelli che dice di voler perseguire, creando quindi una sorta di effetto *boomerang*. Sappiamo tutti che il risultato che di fatto avrà il provvedimento sarà quello di aumentare gli irregolari nel nostro Paese e sappiamo tutti che, con l'aumento delle presenze illegali nel nostro Paese, aumenterà anche l'insicurezza. Siamo quindi di fronte al paradosso di un decreto-legge che si richiama alla sicurezza e che finirà, se approvato così come oggi è scritto, per produrre insicurezza.

del flusso migratorio, che investe il nostro ed altri Paesi. Bisognerebbe davvero fare alleanze, come ha ricordato il senatore Pittella, per arrivare alla possibilità di riformare il Regolamento di Dublino, bisognerebbe non essere isolati in sede di Unione europea, bisognerebbe fare tutto il possibile per stringere rapporti che ci consentano di effettuare veramente dei rimpatri, bisognerebbe fare intese giuste per arrivare alla redistribuzione. Da questo punto di vista, il nostro Governo sta commettendo molti errori e la discussione di questa questione pregiudiziale è un'ulteriore occasione per segnalarli e per invitare la maggioranza ad un ravvedimento, perché se davvero vogliamo avere più sicurezza, nel rispetto dei principi costituzionali e di umanità, bisogna seguire una strada tutta diversa da quella che con il provvedimento in esame si è deciso di imboccare. apre una nuova finestra"). Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno.

vorrei invitare a una riflessione tutti voi, in relazione a un ragionamento che mi sembra oggettivo. Noi stiamo discutendo un provvedimento che di fatto è un provvedimento manifesto.

che si propone di garantire maggiore sicurezza. Come è stato detto da chi mi ha preceduto, il risultato è abbastanza evidente: produrre ulteriore clandestinità e maggiore insicurezza. L'ideologia che sta dietro a questo provvedimento è però molto preoccupante. Esistono dei principi costituzionali e giuridici in questo Paese, non solo nella Costituzione, ma anche prima della Costituzione, che con questo provvedimento si vanno a stracciare. In primo non esiste nessuna emergenza. Ormai questo, prendendo come riferimento il Ministro dell'interno, è dichiarato dallo stesso Ministro: c'è una c'è una riduzione di oltre l'80 per cento degli sbarchi e degli arrivi. Non c'è emergenza e il decreto-legge è uno strumento inappropriato per affrontare la questione. In secondo sulla cittadinanza si stanno introducendo due criteri diversi: il cittadino che per nascita ha la cittadinanza e che commette reati avrà un percorso; il cittadino acquisito e che ha acquisito la cittadinanza avrà un altro percorso. Questo è chiaramente incostituzionale e mette in discussione un principio giuridico fondamentale.

io vi prego, riflettete rispetto a questa pregiudiziale, ma soprattutto riflettete prima di approvare un provvedimento di questo tipo, che apre le porte a un modo di ragionare molto pericoloso in questo Paese e che, come è stato detto, è già stato praticato in questo Paese, con le leggi razziali e con altri provvedimenti di un lontano Novecento.

come il Daspo per chi è ammalato, sono provvedimenti che possono raccogliere applausi demagogici da parte di qualcuno, ma che fanno male a questo Paese. Vado avanti. Vedo che continuate a bombardare l'unico sistema di accoglienza che ha funzionato, che è quello dello SPRAR. Non c'è solo Riace, ma c'è anche un lavoro fatto dai Comuni. Voi lo bombardate, lo mettete in discussione e costruite un sistema emergenziale, anche questo fuori dalle regole della Costituzione, che fa fa sì che possiate trattenere, non si capisce bene dove, per centottanta giorni una persona. Ma riflettiamoci. È questa la strada? Non c'è l'emergenza, allora vi chiedo: qual è una scelta fondamentale che dovreste fare? Lo dico prima di tutto ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, che guardo sempre con molta attenzione: non c'è dubbio che una delle ragioni della crescita della clandestinità in questo Paese sia la legge Bossi-Fini. sono infatti migliaia di persone che accudiscono i nostri padri e le nostre madri che sono in clandestinità per quella legge se non ci fossero loro ad accudire i nostri padri e le nostre madri. Peraltro, con i provvedimenti che state adottando, non so dove andrebbe a finire il *welfare*. Rifletteteci; ragionateci. Non sono la demagogia e la propaganda che possono far affrontare con umanità, legalità e trasparenza il tema dell'immigrazione, ma un ragionamento più serio, meno propagandistico, alla ricerca della verità e non degli applausi e della degli applausi e della facile raccolta di consensi. Io vengo da una Regione dove alcuni anni fa, in molti Comuni

In quegli anni (parlo di cinque o sei anni fa), quegli immigrati erano integrati, lavoravano, stavano dentro a un meccanismo. Spingere sulla paura e sulla pancia produrrà gravissimi danni anche per la sicurezza in questo Paese. Rifletteteci.

Fratelli d'Italia voterà contro queste questioni pregiudiziali perché, se il decreto sicurezza proposto dal Governo ha un difetto, è quello di essere molto fumo e poco arrosto. Non c'è nessun pericolo per la Costituzione italiana, semmai, c'è un pericolo per i cittadini italiani, che non sono adeguatamente tutelati da questo decreto-legge. Noi ci impegneremo in quest'Aula perché questo provvedimento sia all'altezza delle promesse fatte in campagna elettorale dalle forze politiche che oggi governano e con questo decreto buttano fumo negli occhi agli italiani, promettendo, ad esempio, di abrogare la norma (anomalia tutta italiana) della protezione umanitaria, salvo poi inserire in questo stesso testo tutta una serie di eccezioni che rendono del tutto inutile questa finta abrogazione, dimenticando ancora una volta che il Consiglio europeo del 28 e del 29 giugno ha decretato che chi entra illegalmente in uno Stato membro dell'Unione europea deve essere trattenuto. Ma quali norme liberticide, colleghi della sinistra? In Germania il trattenimento di chi entra illegalmente nello Stato tedesco o di chi vi viene trovato oggi è previsto fino a mesi, non fino a sei mesi come vuol fare questo decreto-legge. Ancora, in questo decreto-legge ci dovrebbe essere un principio sacrosanto, che purtroppo non c'è, e cioè che chi si vuole affidare allo Stato italiano per essere protetto deve rispettarne le regole, comprese le regole che disciplinano l'ingresso degli stranieri in Italia. Egregi Egregi signori del Governo, in questo decreto-legge dovete prevedere che la domanda di asilo vada presentata soltanto nel momento in cui lo straniero vuole entrare in Italia, alla frontiera,

l'espulsione immediata per i cittadini dell'Unione europea che stanno sul nostro territorio e sono privi di qualsiasi mezzo di sussistenza. Questo avviene nella civile e democratica Germania e non avviene in Italia e anche su questo il vostro decreto-legge non dice nulla.

dimenticati i reati gravissimi come il furto in abitazione, che desta un grandissimo allarme, il furto con strappo, ma soprattutto, viene dimenticata l'istigazione a delinquere. In particolare, si dimentica di imporre agli imam che predicano sul territorio nazionale di farlo in lingua italiana: troppo spesso l'uso di un'altra lingua e

una clausola di preferenza per gli italiani che stanno all'estero e che vogliono rientrare in Italia. La sinistra dice che ci servono gli immigrati perché gli immigrati di oggi pagano le pensioni degli italiani. C'è da chiedersi, semmai,

che vogliono venire in Italia? Non sarà più facile integrare questi nostri connazionali di origine italiana rispetto ai nigeriani o a tutti coloro che vengono dall'Africa subsahariana? E ancora,

prevedere un vero decreto sicurezza. Perché non prevedete l'abrogazione dell'articolo del codice penale che ha istituito il reato di tortura? Parliamo di una vera spada di Damocle sugli operatori della giustizia,

in colui che stanno per arrestare, vengono accusati addirittura di tortura: basta un turbamento psichico, pensate un po' a cosa siete riusciti ad arrivare, colleghi della sinistra, nella scorsa legislatura. cari colleghi, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà contro questa pregiudiziale perché vuole davvero che quest'Aula si occupi di questi temi e dia una risposta urgente e indifferibile alla domanda di sicurezza del popolo italiano.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono mesi che il Ministro dell'interno alza i toni nel Paese e fa crescere le aspettative degli italiani intorno ai temi di questo decreto-legge. Sono mesi che lo sentiamo promettere il pugno di ferro su sicurezza, immigrazione, rimpatri, come se i due temi fossero perfettamente sovrapponibili o comunque due facce di una stessa medaglia, come se il nodo della sicurezza delle nostre città e delle nostre comunità dipendesse esclusivamente dal numero di immigrati presenti sul nostro territorio e come se, viceversa, una moderna democrazia come l'Italia, nella posizione geografica che occupa, potesse oggi decidere da sola di fare a meno di un fenomeno globale come l'immigrazione o potesse quanto meno decidere di fermare - per fare un esempio concreto - il vento con le mani. Sono mesi che il vice *premier* Salvini ci spiega che quello dei flussi migratori è un problema soltanto di ordine pubblico e di stretta sul respingimento di chi arriva e sul rimpatrio di chi già c'è. Tutto questo decreto-legge è stato scritto in questa cornice. Non è un caso che nel titolo non compaia nessun'altra delle molteplici materie su cui interviene. Avrebbe, infatti, agli occhi dell'opinione pubblica, diluito l'equazione immigrazione uguale insicurezza, su cui la propaganda leghista prova a costruire ormai con ogni evidenza da tanto tempo il proprio consenso. L'intenzione era quella di gettare benzina per giustificare un'emergenza migranti ben al di là della realtà ed è la ragione per cui è stato usato lo strumento del decreto-legge, che richiederebbe presupposti di necessità e urgenza, quando invece, almeno nelle soluzioni prospettate, non si rileva nessuno di questi caratteri. Si tratta, com'è chiaro, di interventi strutturali che modificano discipline di intere materie. Per un verso, si riorganizza la disciplina a tutela dei richiedenti asilo, per un altro si interviene sull'organizzazione dell'Agenzia dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Tra l'altro, su questa materia, si modifica in modo pericoloso il codice antimafia, prevedendo la possibilità di vendere beni confiscati al miglior offerente. Si abbandona, cioè, il principio, seguito in questi anni, per cui i beni sottratti dalla mafia alla comunità debbano tornare alla comunità, con una funzione sociale certa. In più, dietro la logica della privatizzazione, c'è il rischio concreto che il loro acquisto sia effettuato da imprenditori e faccendieri che si muovono in una zona grigia sul confine della legalità. Ho preso due esempi significativi, quello della protezione internazionale e quello dell'Agenzia, per dire quanto poco i singoli contenuti del decreto-legge abbiano da un lato il carattere della straordinarietà e urgenza, dall'altro quello dell'omogeneità, elementi che, come sappiamo, secondo l'articolo 77, secondo comma della nostra Costituzione, sono necessari per legittimare l'esercizio del potere legislativo da parte del Governo. Ma passino anche questi *escamotage* per mantenere alto il clima da campagna elettorale permanente. Ci stiamo abituando a capire che la propaganda è l'ossigeno vero di questa coalizione di Governo. Quello che è preoccupate, però, è la pretesa del Governo di affrontare il tema delle migrazioni come se fossero un fatto emergenziale. È la dimostrazione più plastica che non si è capito nulla di un fenomeno che accompagnerà le nostre democrazie non per anni, ma per decenni. Mettere la testa sotto la sabbia, non vedere che quello che ha avvicinato i continenti ha anche accelerato il ritmo delle migrazioni, pensare di poter scansare i flussi, tutto questo significa soltanto mettere paura al presente usando il futuro e l'Italia invece ha bisogno di quelle opportunità, ha bisogno che il fenomeno migratorio venga governato con scelte che spingano oltre le convenienze immediate e guardino con sapienza e lungimiranza al futuro. Il problema vero è dato dal merito di questo decreto-legge. C'è una cosa su cui il vice *premier* Salvini dice il vero: questo provvedimento da lui fortemente voluto riguarda effettivamente tutti gli italiani. Li riguarda però, purtroppo, perché li colpisce e li colpirà in maniera negativa in un domani non troppo lontano. Il titolo di questo decreto-legge sarebbe dovuto essere, più chiaramente, decreto propaganda e insicurezza, perché questo contiene: o risposte che non sono soluzioni o risposte che sono soluzioni radicalmente sbagliate, che avranno solo l'effetto di rendere meno sicuri tutti gli italiani. Da un lato ci sono le operazioni di distrazione, si cambiano parole per cose che di fatto restano uguali: viene eliminato il permesso di soggiorno per motivi umanitari e lo si sostituisce con permessi con permessi speciali che però di fatto ricalcano quanto già succede oggi. Anche la loro durata sarà la stessa di quella prevista oggi nella maggior parte dei casi. L'unica conseguenza sarà, semmai, così noi avremo uno strumento in meno per dare attuazione al diritto di asilo sancito dalla Costituzione all'articolo 10, un diritto che, come è stato ribadito dalla Corte costituzionale, non è del tutto incasellabile in una tipizzazione rigida. Dall'altro poi ci sono le soluzioni invece radicalmente sbagliate. Se infatti il Governo decide di abbattere gli strumenti di integrazione migliori che il nostro Paese si è dato nel tempo, strumenti che anche con fatica e difficoltà si erano diffusi tra i Comuni e le amministrazioni territoriali, a subirne le conseguenze sarà il livello di sicurezza e di controllo dei nostri territori. La stretta che viene disposta sulla revoca della protezione internazionale e sulla sospensione della domanda di asilo non produrrà espulsioni più semplici. Avremo l'effetto opposto, quello di aumentare la clandestinità e la marginalità. Colui al quale verrà revocata la protezione, non potendo fare ritorno al suo Paese, finirà per restare in Italia, soltanto lo farà da irregolare, da uomo invisibile. Diventerà clandestino anche colui al quale sarà sospesa la domanda di asilo per una condanna in primo grado di giudizio. Oggi la sospensione scatta dopo condanna definitiva, domani, con questo decreto-legge, il principio di non colpevolezza, che vale senza discussione per i cittadini italiani, segnerà per i richiedenti asilo un'eccezione palesemente ai limiti della costituzionalità. Così come per quello che riguarda il periodo di trattenimento presso i centri di permanenza, che viene raddoppiato senza motivo, aumentando così il pericolo concreto che si verifichino abusi e arbitri ai danni dei migranti. Attenzione perché una misura del genere, a così forte impatto sulla libertà personale, rischia di essere in palese contrasto con la Costituzione e con la Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Ancora di più visto che l'unica motivazione alla base sembra essere l'intento punitivo nei confronti dei migranti. Ecco, valutando tutte queste misure, l'unica cosa che grazie a questo decreto-legge risulterà più semplice per i migranti sarà invece uscire dalla legalità e gonfiare così il bacino di persone disperate soggette al richiamo e al ricatto della delinquenza. Eccolo il vostro decreto sicurezza. Da un Governo come quello attuale, che ha messo l'immigrazione in cima alla lista delle sue priorità, ci saremmo francamente aspettati qualcosa di più; di sicuro qualcosa di diverso da questo. Se c'è un aspetto delle politiche repressive che è specifico del fenomeno migratorio, questo poi è la lotta contro le organizzazioni criminali che speculano su situazioni disperate di persone allo stremo delle speranze di vita. In questo decreto-legge però di misure contro gli scafisti, contro il traffico di esseri umani, contro quelli che approfittano e speculano su situazioni di emergenza e di bisogno, non c'è traccia. Il Governo aveva annunciato il pugno di ferro contro l'illegalità e però, poi, non fa nulla in questo decreto-legge per rafforzare la lotta contro coloro che quella illegalità la producono ogni giorno e sopra di essa speculano e si arricchiscono. Dite di voler potenziare i centri per i rimpatri e stanziate 500.000 euro per il 2018 e un milione e mezzo per il 2019-2020; sono briciole che produrranno una diminuzione di rimpatri, anziché un aumento, dato che da quando si è insediato questo Governo si è anche persa di vista una seria ed efficace azione diplomatica, la sola che, come è stato fatto in passato, può consentire ad un Paese come l'Italia di rimpatriare i migranti irregolari nei Paesi di provenienza. L'unica politica estera portata avanti dal vice *premier* Salvini è stata quella con i Paesi che hanno interesse ad indebolire le politiche di integrazione europea e lasciare l'Italia dunque più esposta e più sola nel dibattito, dibattito, come abbiamo detto stamattina. Con questo provvedimento insomma, signor Presidente, il Governo perde la sfida della sicurezza, la perde per l'inefficacia delle risposte che offre, ma la perde soprattutto perché rinuncia all'unica scommessa su cui oggi ha senso investire, quella dell'integrazione. Viene distrutto, come è stato detto, il sistema di accoglienza diffusa per i richiedenti asilo. È uno strumento che in questi anni si era diffuso ed era stato apprezzato dai Comuni perché si basava su un principio semplice, quello per cui è più facile integrare se i numeri ingenti sono distribuiti sul territorio, se viene favorita la fiducia tra chi accoglie e chi è accolto, se chi è accolto entra a far parte di un progetto sociale conosciuto e condiviso. Il Governo ha deciso di non giocare proprio questa partita, preferendo puntare tutto sui grandi centri di accoglienza, con una grande concentrazione di persone, un peggioramento della vita interna e con aumento così delle esigenze di controlli. Verrebbe da chiedersi perché, se non sapessimo che alimentare sicurezza e diffidenza sociale è l'unica strategia che questo Governo sa mettere in campo. È una strada miope, cinica e irresponsabile che questo provvedimento conferma. Insomma, vi siete impegnati e ce l'avete fatta; avete dato con questo provvedimento il peggio di voi stessi, generato aspettative che voi stessi avete alimentato fomentando un clima di paura e di intolleranza, per poi costruire finte soluzioni che, però, invece di migliorare, peggiorano notevolmente le condizioni esistenti, generando marginalità, esclusione ed insicurezza. Il tutto per un po' di propaganda a buon mercato e per distogliere l'attenzione dal baratro nel quale state

È iscritto a parlare il senatore Stefano. Ne ha facoltà. Signor Presidente, il nostro Gruppo non condivide le questioni e le contestazioni di costituzionalità sul decreto-legge. Siamo consapevoli della complessità della discussione in materie quali l'espulsione o la cittadinanza, perché c'è sempre stato un contrasto tra le esigenze di sicurezza, largamente avvertite nel Paese, e i profili giuridici che spesso hanno portato a discussioni molto sottili e complesse. Tuttavia, di fronte al tema del terrorismo jihadista e fondamentalista, il problema della cittadinanza va valutato con realismo perché non si può considerare cittadino meritevole chi ha comportamenti di un certo tipo. Abbiamo visto, del resto, come i fenomeni di integrazione non abbiano risolto le questioni. A volte si è detto che l'emarginazione dell'immigrato spinge verso il fondamentalismo. Non è stato così

di fronte a questi temi, la discussione è indubbiamente delicata e si potrebbe estendere anche a cittadini nati qui da generazioni, quindi semmai il tema della scelta di revocare la cittadinanza a nostro avviso, va esaminato con attenzione. Ne discuteremo nel merito. Le audizioni che ci sono state hanno sollevato problemi complessi di ordine costituzionale però, ripeto, noi abbiamo una realtà contemporanea molto modificata con comportamenti che erano inimmaginabili. Poi si dirà che allora il tema dovrebbe riguardare anche gli italiani che hanno compiuto delitti efferati come sciogliere i bambini nell'acido. Credo che sarebbe legittimo anche in quei casi porsi il problema della cittadinanza perché nessuno di noi si sente concittadino di Brusca o di altri personaggi che poi, semmai, legislazioni premiali hanno eretto

Ci accingiamo a fare un esame di merito del provvedimento. Proprio poc'anzi, con alcuni colleghi, esaminando le proposte di legge di tanti colleghi del Gruppo Forza Italia, abbiamo colto un'attività emendativa intensa che porteremo che porteremo avanti perché ci preoccupa soprattutto la sicurezza sul territorio e la mancanza di personale. Siamo preoccupati per i titoli che ci sono in questo decreto-legge, senza lo svolgimento del tema perché questo è il problema. Ci sono alcuni annunci, alcune affermazioni, che è tipico di questo Governo: avete fatto numerosi annunci, alcuni anche contraddittori e alcuni che dobbiamo ancora capire - parlo della parte economica - ma ne parleremo più in là perché non abbiamo ancora compreso gli annunci sulle pensioni, i redditi, le cittadinanze, se 9 miliardi diviso 9.000 euro fa un milione o fa 6 milioni e mezzo, come teorizzano alcuni novelli economisti

Ad esempio, oggi, colleghi, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Giovanni Nistri, ha svolto un'audizione presso le Commissioni congiunte difesa di Camera e Senato. Diversi colleghi di vari Gruppi hanno partecipato e Giovanni Nistri ci ha detto, parlando dei Carabinieri - ma lo stesso discorso vale per la Polizia o per i Vigili del fuoco - che sono 93.000, hanno un certo numero di persone che andranno presto

si vorrebbe un commissariato più dotato. Leggiamo anche, in questi giorni, la fatica che fa il Governo: aumentiamo a Roma, riduciamo da un'altra parte, non è vero. Insomma: si fa quel che si può con la coperta corta. Oggi il generale Nistri ci ha detto in un'audizione formale o non garantiranno una serie di presidi. Lo ha detto in maniera garbata e rispettosa del Parlamento e delle istituzioni. Ora noi non vediamo queste assunzioni. Colleghi del Governo, non ci sono state durante l'estate perché il ministro Tria non ha firmato la richiesta che lodevolmente il ministro Salvini aveva fatto. In questo decreto-legge ci direte, quando noi le proporremo, che non è questa La sede è la legge di stabilità. Si parlava di un miliardo e questa mattina sui giornali ho letto di mezzo miliardo. Tra mezzo miliardo e un miliardo,

Attenzione a non fare confusione: non mettete un prefetto al telegiornale e un giornalista ai servizi segreti, nel caso in cui i foglietti a Palazzo Chigi noi non voteremo queste pregiudiziali. Daremo un contributo di merito sul decreto-legge perché ci servono strumenti. Penso alla Polizia penitenziaria e alle assunzioni, che vanno decise subito. Per le coperture non c'è problema; si trovano per tutto. Se si deve sforare il *deficit*, lo si faccia per assumere poliziotti, carabinieri e finanzieri.

positiva e propositiva di aggiunta di norme che chiederemo anche sui temi dell'immigrazione, del rafforzamento della polizia locale, degli organici delle Forze di polizia, sugli armamenti e sulle attrezzature tecnologiche e anche sulla parte di natura penale. Vi faremo sicuramente un po' di concorrenza, ma al servizio dei cittadini. Non ci presteremo al blocco di questo decreto-legge, ma non lo prenderemo a scatola chiusa, perché i titoli non ci accontentano, vogliamo la sostanza!

tende ad allontanarsi dal merito dell'ordine del giorno e dagli argomenti in discussione, mi permetto di cercare di ricondurre la discussione al merito del voto sulle pregiudiziali ricordando che, se si volge lo sguardo al passato anche di recente espressione, è possibile notare che in più occasioni il legislatore ha fatto ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza al fine di disciplinare materie affini a quella di cui oggi si discute. Si pensi che, tra la fine della XII e l'inizio della XIII legislatura, si registra una catena di sei decreti-legge recanti disposizioni urgenti in materia di politica di immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea. È evidente, quindi, che il Governo, nel corretto esercizio della funzione legislativa che gli è propria, non travalica le attribuzioni costituzionalmente garantite ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione andando a intervenire in materie coperte da riserva di legge, alla quale è riconducibile anche lo strumento del decreto-legge. Ciò senza considerare il nesso funzionale esistente tra il decreto-legge e la legge di conversione che, lungi dal sanare eventuali vizi del decreto-legge (che noi non intravediamo), ne garantisce comunque lo sviluppo giuridico e politico. Come precisato anche dalla Corte costituzionale, le ragioni di economia procedimentale giustificano l'esistenza di questo procedimento legislativo bipartito tra un provvedimento del Governo e una sua successiva conversione in sede parlamentare. Rispetto poi al merito delle molte cose dette negli ultimi interventi, ci sarà l'opportunità, in sede di discussione del in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge, di sviluppare alcuni argomenti che sono stati toccati in queste dichiarazioni: molti di questi non ci convincono, ma lo sosterremo nella sede opportuna, che è quella, appunto, del dibattito parlamentare sul disegno di legge di conversione. Per questo motivo il MoVimento 5 Stelle voterà contro le proposte di

Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, membri del Governo, il documento che esaminiamo riguarda la proposta, comunicata alla Presidenza il 5 luglio scorso, di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. Nel corso della XVII legislatura questa Commissione era già stata istituita e - come si evince dalla relazione conclusiva, approvata nel mese di febbraio 2018 ha svolto un'attività significativa di audizioni e indagini sulle reali dimensioni del fenomeno allo scopo di arrivare a una ricostruzione e valutazione del quadro normativo e della tutela giurisdizionale. Tuttavia, essere qui oggi, 16 ottobre 2018, e parlare ancora una volta di istituire una Commissione di inchiesta per approfondire le reali dimensioni del fenomeno femminicidio mi pone nella condizione di riflettere su un principio:

non è solo l'atto di uccidere una donna, ma è il termine comprensivo di tutti i soprusi che una donna può subire durante la propria vita.

Sono convinta che, per approfondire le reali dimensioni del fenomeno, bisogna partire proprio da questa riflessione, semplice all'apparenza, ma piena di contenuti, se prescindiamo dalla considerazione del fenomeno come aggressione fisica di un uomo contro una donna e includiamo nel nostro esame tutte le vessazioni, a livello psicologico, socioeconomico, minatorio, vessatorio e sessuale. Non posso però esimermi dal soffermarmi brevemente sugli interventi legislativi in materia e, in particolare, sottolineare l'importanza che ha assunto a livello mondiale la Convenzione di Istanbul del 2011, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante in materia di protezione dei diritti della donna contro ogni forma di violenza. A differenza di ogni altro intervento normativo in materia, la Convenzione ha riconosciuto in modo palese che l'elemento fondamentale per prevenire la violenza contro le donne è il raggiungimento dell'uguaglianza di genere, di fatto e di diritto. Nella Convenzione si legge infatti quanto segue: «con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata». In seguito al riconoscimento della Convenzione nel 2013, il Governo è intervenuto con un decreto‑legge, poi convertito in legge, che ha introdotto nel diritto penale sostanziale e processuale misure volte a contrastare la violenza di genere e la previsione di un piano straordinario di azione per dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione e repressione contenute nella Convenzione stessa. È stata così riconosciuta giuridicamente la violenza domestica che viene agita prevalentemente dagli uomini contro le donne, soprattutto fra le mura domestiche, proprio nell'ambito ritenuto più sicuro, e nella cui definizione sono compresi molteplici azioni e comportamenti che mirano tutti all'affermazione del potere e del controllo sull'altra persona, sul suo agire e pensare. Questo tipo di violenza è spesso direttamente collegato al concetto di violenza assistita, anch'essa riconosciuta dalla legge, riferita soprattutto ai minori costretti ad assistere, facendo quindi esperienza di qualsiasi forma di maltrattamento, a episodi di violenza in danno di figure familiari di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte e minori. Relativamente, poi, all'attenzione specifica di questa Commissione per il femminicidio, non mi dilungo, sembrandomi esaustiva la definizione del termine data dall'antropologa Marcela Lagarde: «La forma estrema di violenza di genere contro le donne, prodotto dalla violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato, attraverso varie condotte misogine poste in essere tanto a livello sociale, quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in una posizione indifesa e di rischio, possono culminare con l'uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa». Oggi la violenza di genere è studiata e analizzata rispetto ai suoi vari aspetti sociali, antropologici e culturali che hanno grande rilievo, anche in ogni branca delle scienze umane, della psicologia, della letteratura e della politica, mettendo in luce la diversità della materia con l'eterogeneità non solo di di rapporti personali e familiari, ma anche di diversa visione del mondo. Tuttavia, da qualunque angolazione si guardi si evince che oggi questo fenomeno costituisce una vera emergenza sociale e culturale che non conosce confini geografici, distinzioni di cultura, differenze e *status* sociali. Tutto ciò premesso, passo a elencare l'articolato del provvedimento oggi in discussione per l'istituzione della Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. L'istituzione viene prevista all'articolo 1 con specifica attenzione al femminicidio. La durata della Commissione è di un anno dall'insediamento dell'Ufficio di Presidenza. Tale durata è motivata dalla finalità di questa instauranda Commissione di consolidare l'attività svolta durante la passata legislatura. Avendo infatti la Commissione precedente svolto ampia attività di audizioni e indagini conoscitive del fenomeno, ora è giusto lavorare in modo più specifico al fine di individuare in maniera puntuale le modifiche e soprattutto le innovazioni normative eventualmente da apportare a quanto esiste già e meccanismi più rapidi dal punto di vista burocratico per un'adeguata prevenzione del fenomeno. In ordine alla ridotta durata è stato modificato anche il comma 5 dell'articolo 6 sulle spese di funzionamento della Commissione. L'articolo 2 attiene ai compiti e alle funzioni della Commissione, che deve svolgere indagini, accertamenti, verifiche, ponendo particolare attenzione ai progetti educativi che vengono svolti nelle scuole di ogni ordine e grado proprio per far crescere una vera cultura della prevenzione e dell'accettazione e valorizzazione di ogni diversità, a cominciare da quella di genere. Penso che, però, proprio nella lettera *i)* dell'articolo 2 stia il vero obiettivo dei lavori della Commissione parlamentare: proporre interventi normativi. A volte basterebbe anche solo applicare le leggi esistenti o adoperare il buonsenso perché, proprio per la peculiarità del fenomeno in cui è vero che esistono vittime dirette delle azioni di violenza, sarebbe opportuno allargare lo sguardo e pensare a nuovi strumenti che non consistano solo in modalità e misure repressive nei confronti di chi commette le violenze, relegando così la gravità del fenomeno a un atto di violenza qualsiasi, quasi sminuendone la gravità stessa, pensando di aver raggiunto il fine di ottenere giustizia unicamente al momento dell'irrogazione della pena per il reato commesso. Occorrerebbe pensare a misure che prevedano anche e soprattutto una metodologia di prevenzione, di accompagnamento psicologico, di riabilitazione. Invero, è opportuno realizzare un'adeguata rete di prevenzione e un efficace contrasto a ogni forma di violenza di genere attraverso una revisione concreta del piano d'azione straordinario già previsto, consentendo l'organizzazione di percorsi strutturati nonché una più equa distribuzione dei fondi e delle risorse economiche tra le strutture esistenti, tenendo conto anche delle specificità delle stesse e dei bisogni delle vittime, basandosi sulle buone pratiche già realizzate a livello territoriale, anche grazie ad azioni di soggetti privati. Tutto ciò senza dimenticare che lo Stato deve essere il soggetto più impegnato in ogni azione. Concludo questo mio intervento con l'auspicio che ognuno di noi, al di là del proprio impegno in Commissione, in Parlamento, e della propria attenzione verso il fenomeno del femminicidio e della violenza in ogni sua modalità, voglia farsi garante di: promuovere una cultura che non discrimini le donne, prevenire la violenza maschile sulle donne, proteggere tutte tutte le vittime di violenza, punire, cioè perseguire i crimini, procurare indennizzo e risarcimento, non solo in termini economici ma anche in termini di assistenza morale e psicologica. Infine, se mi permettete, voglio rivolgermi a tutte le donne, facendo mie, affinché siano di monito, le parole di Rita Levi Montalcini: «Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza».

Prego pur anticipando il voto favorevole del mio Gruppo su questo articolo, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulle perplessità che ci suscita la limitazione temporale prevista dall'emendamento della relatrice. La riduzione della durata dell'attività della Commissione di inchiesta a un solo anno, a decorrere dal suo insediamento, non potrà di fatto consentire il pieno svolgimento di un'indagine approfondita sulle reali dimensioni né sulle cause del fenomeno, e renderà più difficile mettere in luce tutte le informazioni necessarie per proporre soluzioni idonee a rafforzare norme di carattere preventivo e di contrasto. Quindi, sarebbe stato per noi più opportuno non modificare il testo originario dell'articolo 1 che prevedeva che la durata in carica della Commissione fosse coincidente con quella della legislatura. solo pochi giorni fa a vincere il premio Nobel per la pace sono stati una giovane attivista yazida, che, rapita nel 2014 dall'ISIS, dopo tre mesi di sequestro è riuscita a scappare e da allora con la forza e il coraggio delle parole racconta al mondo le violenze subite, e, con lei, un medico congolese diventato nel suo Paese uno dei maggiori esperti mondiali nel trattamento dei danni fisici dovuti agli abusi sessuali. Sarebbe difficile per la nostra discussione oggi non partire da qui, dal significato e dalla forza di questo importante riconoscimento. Un riconoscimento che racconta molto di quanto la violenza sulle donne oggi rappresenti uno dei più atroci e insopportabili atti di sopraffazione e di guerra di un essere umano su un altro essere umano, di quanto in quei gesti vi sia la ricerca aberrante e distruttiva dell'affermazione di un potere, di un dominio, di un pezzo di umanità sopra un altro pezzo di umanità, di un genere su un altro genere. Nella precedente legislatura

abbiamo anche deciso di dotarci di una Commissione perché era necessario che gli strumenti messi in campo fossero verificati e sondati, nella consapevolezza che troppo poco ancora emerge rispetto a quanto si consuma ogni giorno. Consapevoli dunque della parzialità del lavoro, scegliemmo di dar vita a una Commissione parlamentare monocamerale d'inchiesta sul femminicidio, perché rigore, serietà, responsabilità - che sono per loro natura lontani da propaganda, promesse e annunci impongono dubbi non certezze, impongono una verifica costante del lavoro fatto e dell'efficacia degli strumenti individuati. Era evidente che questo lavoro non poteva essere chiuso rapidamente, per quanto condotto anche nel modo migliore possibile. Per questo abbiamo ripresentato e avanzato la proposta di mettere nuovamente in piedi la Commissione all'interno e siamo stati felici che alla nostra proposta si siano aggiunte quelle di tante altre forze politiche, di maggioranza e non. Per questo però ci sorprende e, al contempo, ci delude la scelta di mantenere in vita la Commissione solo per un anno, di farla nascere con una scadenza tanto ravvicinata. Gli stessi che la volta scorsa ci accusavano che per farla funzionare in maniera adeguata il tempo fosse poco (mi riferisco ad esempio ai parlamentari della Lega) oggi sostengono l'inutilità di tempi così lunghi. Questa volta si tratta di un fenomeno troppo delicato per speculare; si tratta di un fenomeno drammatico per fare propaganda e vi chiediamo davvero di non farla anche su questo. Per noi la scelta giusta era far andare avanti la Commissione per l'intera legislatura. Invece voi ci mettete di fronte a un'altra scelta: un anno di lavoro, una Commissione a scadenza. Siamo certi che per il lavoro da fare, per le verifiche da effettuare, per i dati ancora da raccogliere, per le cose da realizzare non sarà sufficiente. Siamo certi, però, che la scelta di ripartire dal lavoro già fatto dalla precedente Commissione ci aiuterà e ci consegnerà un buon punto di partenza, ma ovviamente per noi non potrà essere sufficiente. Ciononostante, nella convinzione che sempre, e in particolare su un argomento di questo tipo, il meglio è nemico del bene, per oggi diciamo meglio questo che niente, confidando nel fatto che tra un anno, se ve ne dovesse essere ancora l'esigenza, lascerete da parte logiche di battaglia o di speculazione politica e sceglierete pensando unicamente all'interesse di quelle donne - purtroppo tante - che ci chiedono ancora aiuto, che ci chiedono di non girarci mai dall'altra parte; che chiedono alla politica che la violenza sulle loro vite, sui loro corpi, finisca di essere un fatto privato per diventare finalmente un fatto pubblico, arrivando così ad investire le nostre coscienze e a imporci la necessità di rafforzare su questo terreno una battaglia che è, sopra ogni altra cosa, una battaglia culturale, civile e sociale.

condividiamo i principi della nostra Costituzione circa l'assenza di distinzioni di razza, di religione e di lingua e tanto più non condividiamo nessun tipo di distinzione.

L'Organizzazione mondiale della sanità ha condotto un esame su 81 Paesi del mondo e ha verificato che il 35 per cento delle donne, nel corso della propria vita, ha subito una qualche forma di violenza: segregazioni, deprivazione, intimidazioni, *stalking*, prostituzione coatta - sentite quanta violenza? - violenza sessuale, mutilazioni genitali, abuso sui minori, violenza assistita,

abbiamo capito che la violenza carnale non è un delitto contro la morale, ma un delitto contro la persona. Abbiamo fatto dei passi importanti dal punto di vista normativo: facciamoli anche dal punto di vista reale. Noi vogliamo questo per l'Italia.

dal proseguimento di quelle indagini sulla reale dimensione e sulle cause del femminicidio avviate nella scorsa legislatura dalla prima Commissione d'inchiesta sul femminicidio. I dati raccolti da quella Commissione, i dati forniti dalle procure, dalle Forze di polizia, ma anche le oltre sentenze analizzate - emesse dal 2012 al 2016 - confermano un dato: le donne, per oltre il 75 per cento dei casi, continuano a morire per mano di uomini in un ambito familiare, nell'ambito che avrebbe dovuto proteggerle maggiormente. Ciò su cui non è stato possibile stilare una precisa statistica nella scorsa legislatura è sul movente: rapporti malati di gelosie ossessive e ossessive sottomissioni, anche per motivi economici. i casi di assoluzione anche per infermità mentale (oltre il 53 per cento delle assoluzioni), mentre le pene inflitte, per oltre vent'anni, non hanno svolto alcuna funzione deterrente, e le donne continuano a morire per mano degli uomini. Uno dei compiti della Commissione Commissione sarà allora quello di andare ad indagare sulle cause, intanto dando la possibilità a queste donne di avere dei luoghi dove denunciare violenze e maltrattamento: centri antiviolenza, Pronto soccorso, Forze dell'ordine, purché con personale prontamente formato ad accogliere e riconoscere i rischi. Le donne, infatti, spesso non denunciano e fanno apparire anche incomprensibili i dati italiani rispetto a quelli del resto dell'Europa. Un problema culturale, dunque, che coinvolge indiscutibilmente indiscutibilmente l'educazione al rispetto, al rispetto degli altri, al riconoscimento della parità dei diritti e dei doveri nella diversità dei ruoli e dei compiti svolti, della complessità e difficoltà per le donne nel conciliare lavoro e cura familiare, non ancora in condizioni di parità. Molto è stato fatto nella scorsa legislatura: l'introduzione della fattispecie di violenza assistita, la remissione della querela solo in fase processuale, le intercettazioni per *stalking*, il gratuito patrocinio delle vittime. di questa Commissione riservare attenzione agli effetti e al monitoraggio della vigente normativa, anche in confronto con le normative europee. Ma mi lasci dire, signor Presidente, che sarà molto importante anche che questa Commissione si occupi della valutazione dell'impatto che le nuove proposte di modifica dell'ordinamento possono produrre, perché la violenza domestica, che spesso precede e annuncia l'omicidio, venga presa in carico dei tribunali al momento della separazione e del divorzio, a tutela della parte offesa, ma soprattutto a tutela e nell'interesse

rispetto al principio stesso di uguaglianza, conquistato con fatica e forse mai ancora completamente attuato; un'uguaglianza che noi chiediamo venga esercitata in coppia, nel matrimonio, tra i coniugi, ancor prima che nel divorzio. Concludo, signor Presidente, sottolineando che affermare la cultura del rispetto

l'articolo 3 è l'articolo del «come»: come dovrà funzionare questa Commissione;

tante reiterate denunce che sono state fatte, dopo i dati drammatici che sono stati evocati più volte in quest'Aula, anche negli ultimi minuti, di un femminicidio ogni tre minuti, è impossibile credere che ancora si creino situazioni di questo tipo e, soprattutto, che la violenza femminile assuma sfumature di una complessità tale da essere presente in tutti gli ambienti sociali, in tutti i contesti culturali, in tutti gli ambiti professionali. Noi eravamo abituati a considerare la violenza come un sottoprodotto culturale. Viceversa, ci rendiamo conto che il violento potrebbe essere - come dire - accanto a noi in qualunque momento, ma non riusciamo a capire come questa violenza possa diventare un oggetto reale di denuncia in tempi che permettano un intervento precoce e quindi evitino la degenerazione, per esempio, del femminicidio. Ma non è solo il femminicidio quello che ci preoccupa. Ci preoccupa, soprattutto, il dilagare di una denuncia costante e continua, che sta creando come una sorta di reazione a valanga. Pertanto, ci rendiamo conto che è violento anche ciò che il Presidente faceva notare pochi minuti fa: il semplice fatto che, quando una collega parla, il livello del brusio dell'Aula rende in qualche modo più difficile identificare la sua voce rende più difficile mettere a fuoco ciò che sta dicendo. Anche questa, ha detto il Presidente, è violenza: è un esempio straordinario della concretezza dei piccoli gesti che, in qualche modo, mortificano il femminile. Altrettanto grave, è stato detto più volte, è la violenza che viene perpetrata a livello economico attraverso la nota discriminazione, in quanto le donne sono pagate il 20 per cento di meno. È innegabile la violenza che viene fatta anche attraverso la selezione delle persone, attraverso il linguaggio sessista che viene utilizzato sui *social media*. Io credo che compito di questa Commissione sarà riuscire a identificare le mille forme della violenza, a partire proprio dalla violenza del quotidiano, per aumentare il livello di sensibilità di tutti noi e per trasformare una Commissione d'inchiesta, non solo in uno strumento di denuncia, ma anche in un'occasione opportuna per modificare comportamenti e per riappropriarci del rispetto della dignità del femminile, che poi altro non è che rispetto della dignità di ognuno di noi.

Signor Presidente, siamo qui a votare l'articolo 4 che stabilisce che la Commissione sia composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione del numero dei componenti dei Gruppi parlamentari ma assicurando anche l'equilibrata rappresentanza dei generi. Quindi, cari colleghi uomini, vi prego di porre la massima attenzione. Io stessa, ascoltando gli altri interventi, ho avuto modo di conoscere aspetti di questo dramma incredibile,

che diventano vittime innocenti di questo fenomeno che ha colpito e colpisce il nostro Paese negli ultimi anni in maniera crescente.

da una linea sottile dalla complicità e non possiamo permettercelo. Per questo dobbiamo alzarci tutti in piedi e dire che non ci stiamo e che siamo tutti dalla stessa parte, uomini e donne. Questa battaglia dobbiamo farla insieme. Insieme, con la stessa intensità e determinazione, possiamo combattere questa battaglia di civiltà, che è culturale e sociale, prima ancora che politica. donne che vengono molestate e umiliate in ambito domestico. Vedete, c'è un'attenzione molto forte alla minaccia esterna, alla minaccia che viene da fuori, da fuori casa o da fuori il Paese. In queste settimane e in questi mesi il

cui la prevaricazione a volte è psicologica per sfociare poi nella violenza fisica e chi la subisce finisce per sentirsi prigioniera, sola, sola, privata della propria libertà, incapace di reagire. Il femminicidio spesso è l'atto ultimo, più tragico di queste vessazioni che sono ripetute. È per tale ragione che questa battaglia la vogliamo fare insieme, uomini e donne, con la convinzione profonda che l'amore vada conquistato, coltivato, custodito e mai - dico mai - rubato.

una ogni cinque giorni, ogni sessanta ore. Sappiamo che i femminicidi avvengono soprattutto nel contesto di una separazione, quando una donna vuole iniziare una nuova vita. Purtroppo la concezione maschilista, secondo la quale la donna è considerata una proprietà, è ancora nella testa di troppi uomini, per i quali una separazione rappresenta una lesione di quell'onore maschile che fino al 1981 trovava copertura in un'infame norma del codice penale, quella che prevede una riduzione della pena nei casi di femminicidio susseguenti ad un tradimento da parte della donna. E allora la domanda da farsi è cosa si deve fare per contrastare il fenomeno. Da una parte, bisogna rafforzare la tutela preventiva introdotta con la legge del 2001, ma che non ha portato ai risultati attesi. Non è accettabile che certe donne che hanno denunciato il *partner* continuino a subirne i comportamenti violenti perché lo Stato non è stato in grado di garantire l'adeguata protezione. I provvedimenti cautelari del non avvicinamento all'ex coniuge e ai figli devono essere controllati meglio e in questo senso il braccialetto elettronico proposto con il decreto sicurezza sarebbe una misura efficiente, ovviamente sempre a condizione che lo Stato se li procuri, dato che oggi mancano dove ce ne è bisogno. In più, i reati di percosse e lesioni personali e di maltrattamento in famiglia devono essere presi più sul serio dalle Forze dell'ordine, perché spesso sono i primi segnali di violenza in una spirale che porta al femminicidio. Non è più tollerabile che a tante donne che decidono di denunciare la violenza venga risposto che devono risolvere il litigio in famiglia. Ci vogliono Forze dell'ordine sensibilizzate e preparate con apposita formazione per contrastare la piaga della violenza contro le donne. La condanna sociale nei confronti di chi commette violenza deve essere assoluta e generalizzata, senza attenuanti di alcun genere e dobbiamo sensibilizzare le donne per una forte presa di consapevolezza della propria autonomia e della propria libertà da ogni forma di sopruso psicologico, materiale o sociale che sia. Solo così le donne troveranno sempre più la forza di denunciare o di prendere le distanze perché sentiranno attorno a sé una rete di protezione e solidarietà sociale, ma soprattutto tutti dobbiamo lavorare per raggiungere una società dove uomini e donne sono sullo stesso livello, perché il femminicidio è il punto estremo di degenerazione di quella odiosa cultura che nega pari opportunità e dignità a uomini e donne. Purtroppo nei posti di potere le donne sono ancora sottorappresentate, la pubblicità le ritrae prevalentemente come oggetto sessuale e per le posizioni importanti nella lingua italiana si fa ancora ricorso al maschile. È anche su questo che bisogna lavorare con norme efficaci, da un lato, e una forte iniziativa culturale, dall'altro. Per questo ben venga questa Commissione e che possa lavorare con decisione per questi obiettivi.

e in altri Paesi, per informare e far capire. Quello che avviene attorno a noi, però, non è un caso, non è il frutto di un *raptus* di follia. Sento ancora qualcuno che pensa che coloro che uccidono la propria *partner* o i figli siano presi soltanto da un *raptus* di follia; non è passione, non è gelosia, non è amore. Questo ancora non è chiaro per la maggior parte dell'opinione pubblica e spesso per i *media*. Sappiamo che alcune parole spiazzano, fanno paura per le consapevolezze che evocano e per le responsabilità che denunciano. Il termine «femminicidio» è una di queste parole, che è nata proprio per indicare che le uccisioni di donne sono fatte in quanto donne. Ragazze uccise dai *partner* o dai padri perché magari rifiutano il matrimonio che viene imposto o il controllo ossessivo sulle loro vite.

Marcela Lagarde, antropologa messicana, sostiene che con la parola «femminicidio» si indica un problema strutturale che va al di là là dell'omicidio e riguarda tutte le forme di discriminazione e violenza di genere che hanno la forza brutale di annullare la donna nella sua identità e nella sua libertà, non solo fisicamente, ma anche nella dimensione psicologica, nella socialità e nella partecipazione alla vita pubblica. Quindi è importante istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, ma non basta.

Con la legge n. 77 del 27 giugno del 2013, l'Italia ha proceduto alla ratifica e all'esecuzione della Convenzione di Istanbul, che il Parlamento la votò all'unanimità. Essa chiedeva agli Stati impegni molto concreti, tra cui proprio il sostegno e il potenziamento dei centri antiviolenza e un'opera di prevenzione attenta, iniziando dalle scuole. Tutti coloro che si sono occupati di violenza maschile sulle donne sanno bene che il fenomeno ha radici culturali profonde e che, per poter intervenire in maniera efficace, è fondamentale iniziare a lavorare con le nuove generazioni, sui bambini e sui ragazzi, su coloro che hanno la possibilità di non far sedimentare su loro stessi pregiudizi e stereotipi di genere, che portano appunto a guasti indelebili nelle relazioni interpersonali. Ecco perché la Convenzione di Istanbul, all'articolo 14, prevede ad esempio l'introduzione di una forma di educazione all'affettività nelle scuole di ogni ordine e grado; una scelta normale, che nel nostro Paese non è stata ancora compiuta. Da anni i centri antiviolenza aspettano il finanziamento del Piano nazionale. Stiamo parlando di cifre con cui a malapena si possono pagare le bollette, eppure nonostante siano pochi euro, nonostante le sollecitazioni delle reti e i continui

nel *dossier* sul femminicidio della Commissione parlamentare d'inchiesta della scorsa legislatura. Sono dati drammatici. Nel 2017 sono state 113 le vittime di femminicidio; nel 2016, in Italia, sono state uccise 115 donne; il 2015 ha visto 120 vittime. Quest'anno i numeri non sembrano essere meno confortanti, così come ogni giorno ci confermano le cronache. è certamente cresciuta anche l'attenzione nei confronti di questa forma così grave di violenza, si sono moltiplicate anche le prese di posizione, le prese di coscienza forti, di donne e di uomini. Occorre però andare più in profondità, occorre anche una cultura dell'ascolto della vittima, a partire dal riconoscimento che il femminicidio, lo *stalking* e i maltrattamenti, oltre alla violenza sessuale, sono forme di violenza di genere, rivolta - appunto - contro le donne in quanto donne. Occorre partire da qui, da quei dati che citavo, per raccogliere altri dati secondo un'ottica di genere, per capire se le donne che chiedono aiuto vengano davvero protette o se, invece, vengano lasciate sole. Spesso mancano i luoghi per accoglierle, i fondi non sono sufficienti, le case rifugio spesso chiudono, oppure le donne non ricevono informazioni esatte, pensano che se denunciano non possono avere protezione perché nessuno magari le ha informate compiutamente dell'esistenza della possibilità degli ordini di allontanamento Quindi bisogna indagare a fondo, bisogna mettere in campo proposte e strumenti che possano aiutare le donne, moltiplicare i centri antiviolenza, introdurre modifiche normative alle leggi esistenti, intervenire per esempio sulla formazione delle Forze dell'ordine e per questo bisogna ancor di più insistere e adoperarsi. Succede anche che mentre noi oggi stiamo per votare

Quindi istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta è assolutamente importante, ma bisogna trovare la strada per svelare fino in fondo tutti gli aspetti di questo problema drammatico e richiamare alla loro responsabilità gli uomini, quelli che hanno ruoli pubblici e ricoprono cariche di prestigio, e le istituzioni. Inutile dire che certamente ci sono stati tanti passi avanti in questi anni. L'attenzione è cresciuta, così come la formazione, anche dal punto vista culturale; certamente c'è stato un atteggiamento diverso di protezione ma ancora abbiamo davvero molto da fare. La strada è lunga e se oggi l'ONU parla di femminicidio anche in relazione all'Italia è perché qui ci sono state donne che per anni hanno reclamato un riconoscimento - anche per le donne in quanto donne - di quei diritti umani affermati a livello universale

Signor Presidente, comincio da qualche dato per ricostruire l'evidenza di un fenomeno che perlopiù resta sommerso. Secondo l'osservatorio Eures, ogni due giorni e mezzo in Italia viene uccisa una donna in ragione del suo essere donna - il che vuol dire una donna ogni sessanta ore - e mentre cala il numero degli omicidi, cresce il numero degli omicidi di donne, i cosiddetti femminicidi, che sono il 36,7 per cento del totale. E ancora - e non sono solo numeri ma persone - nei primi sei mesi del 2018 sono stati denunciati circa 2.600 casi di violenza. Si tratta perlopiù di violenza domestica ma le statistiche ci dicono che sono in crescita anche le violenze di gruppo e che aumenta il numero delle minorenni coinvolte. Ma ogni dato continua a rappresentare la classica punta del classico *iceberg* e infatti anche l'Organizzazione mondiale della sanità conferma che la violenza di genere costituisce una questione strutturale, un fenomeno di dimensioni globali che definisce un flagello, un flagello sociale che rappresenta la prima causa di morte delle donne. Insomma, cari colleghi, è un mondo che attraversa il mondo, una malattia sociale trasversale a tutte le latitudini geografiche, a tutte le appartenenze etniche, a tutti i ceti sociali, alle religioni e all'età. 7 milioni le donne che hanno subito una qualche forma di violenza nella loro vita e negli ultimi dieci anni - lo voglio dire e sottolineare, perché ci si pensa sempre e troppo poco - sono oltre 1.700 gli orfani di femminicidio. Femminicidio è un termine che usiamo e non conosciamo, un neologismo antico - mi piacerebbe dire - entrato di recente nel dizionario linguistico e nel parlare corrente, ma che racconta un male secolare. Per questo parlo di un neologismo antico. È forse una parola nuova, anche se il fenomeno nella storia accade da sempre e ovunque. Perché usiamo una parola nuova? La usiamo per rafforzare un concetto e per articolare il concetto che ci dice dell'uccisione di una donna in ragione del suo essere donna. Per estensione, femminicidio è non solo questo, ma qualsiasi forma di violenza sistematica esercitata sulle donne, di cui l'omicidio rappresenta l'atto estremo, ma che in genere è preceduto da una serie reiterata di condotte violente, in difetto in difetto di una presunta subalternità del genere femminile. Il termine femminicidio - le parole hanno un senso - è una categoria interpretativa perché introduce nella cultura e, in taluni Paesi, anche nel diritto una percezione diversa delle violenze sulle donne. tratta, infatti, di violazioni di diritti umani. Questo è il punto. Ha pensato a chiarirlo la criminologa statunitense Diana Russel, che ha canonizzato questo termine intendendo l'omicidio volontario di donna in quanto donna. È andata ancora più avanti l'antropologa e parlamentare messicana Marcela Lagarde, che ha dato al termine un'interpretazione estensiva, che ha stigmatizzato il concetto e che, addirittura, nel Parlamento messicano non solo ha introdotto una Commissione, come la nostra, d'inchiesta sul femminicidio, ma è arrivata a denunciare quell'aspetto di diritto consuetudinario che fa sì che un omicidio di donna sia meno grave di un omicidio. Sempre Lagarde è riuscita, sulla base anche del lavoro della Commissione, a far introdurre nel codice del Paese il reato di femminicidio o la sua aggravante (una nuova fattispecie e una aggravante). In Europa non esiste in alcun ordinamento questo reato, come non esiste in Italia. Cionondimeno usiamo questo termine, e lo dobbiamo usare con un senso di responsabilità. Molto altro

L'istituzione della Commissione che oggi discutiamo è in linea con un bisogno, con le direttive internazionali e, non da ultimo, con la Convenzione di Istanbul,

per proteggere le donne, per prevenire la violenza domestica e per perseguire i trasgressori, riaffermando quel principio, ormai inserito nel diritto internazionale, della violenza sulle donne come violazione di diritti umani fondamentali. Sono tante le tappe che portano a questa conquista e a questa affermazione. Io ne voglio ricordare soltanto quattro delle tante che potrei. Parto dalla prima, dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 e dall'abolizione dal nostro

1996, frutto di un dibattito parlamentare, durato oltre quindici anni, per arrivare a un'intesa trasversale e per sancire un principio che le giovani forse danno per scontato, ma che scontato non era. Infatti, è soltanto con la legge del 1996 - mio figlio aveva già un anno - che le violenze sessuali sono non più «reati contro la moralità pubblica e il buon costume», ma «reati contro la persona»: una conquista tardiva - direi - in un Paese civile. Ancora, la terza tappa fondamentale la legge n. 38 del 2009, la cosiddetta legge anti-*stalking*, quella legge che va a colmare una lacuna grave e pericolosa, introducendo una nuova fattispecie di reato sulle condotte di persecuzione reiterate. Da ultimo, vi è la legge n. 119 del 2013, che rafforza quanto previsto dalla cosiddetta legge anti-*stalking*, introducendo aggravanti e novità fondamentali. Non entro nel dettaglio normativo, ma la chiamiamo impropriamente «legge anti-femminicidio», quando non lo è, perché non esiste questo reato, ma è una legge che punisce gli autori della violenza. In conclusione, è necessario che si prosegua sul cammino già segnato precedentemente e riteniamo necessario istituire anche in questa legislatura la Commissione d'inchiesta sul femminicidio. E lo riteniamo non solo sulla base che vi ho riferito, ma perché è un'esigenza reale; non si pensi che sia retorica femminile e non si pensi che su materie di questo genere ci possa essere un *copyright* ideologico. È un'esigenza reale, perché esiste un fenomeno strutturale e complesso, con dimensioni quantitative, ma soprattutto con coinvolgimenti qualitativi di vittime e persone. Il Gruppo Fratelli d'Italia voterà

il monitoraggio, che è un aspetto invece molto delicato e controverso, perché in Italia abbiamo delle stime, ma non delle statistiche, e questo aspetto è un *vulnus* della Commissione. Voteremo per la sua istituzione anche se manca, nel quadro delle violenze sulle donne, tutta quella pratica abominevole dell'utero in affitto, che è una pratica di mercificazione sul corpo femminile. *(Applausi dal Gruppo FdI)*. Mi auguro che nell'attività della Commissione si colmi siffatto vuoto e si parli

un fatto individuale, ma è la difesa di un bene comune, dei diritti fondamentali e delle libertà individuali. Questo sì è un impegno che richiama tutti, nessuno escluso, a un'assunzione di responsabilità collettiva e condivisa, nella convinzione che le leggi da sole non bastano, nella convinzione che le Commissioni speciali da sole non bastano, se non sono accompagnate da un cambiamento culturale e di mentalità.

presuppone una capacità di modificazione di un insieme di comportamenti che vanno monitorati, modificati e attuati. Si tratta, cioè, di un terreno che capovolge consuetudini, abitudini culturali e qualità sbagliata di relazioni tra uomini e donne. l'istituzione della Commissione anche in questa legislatura assume un significato estremamente importante. Occorre seguire l'attuazione di tale legge, e non solo perché ci dobbiamo dotare anche dei numeri

Perché abbiamo avuto una perplessità - anche se il Partito Democratico voterà a favore dell'istituzione anche in questa legislatura della Commissione - sul fatto che si è dato un limite alla durata

il femminicidio e ogni forma di violenza e discriminazione verso le donne, ha bisogno di un tragitto lungo, perché questo fenomeno non è emergenziale, ma è strutturale e tocca le radici anche antropologiche di come si sono determinati i rapporti di violenza, la sopraffazione e il possesso dentro le società moderne. Non è un caso che il tema viene affrontato in sede non solo nazionale, ma anche europea

lo *stalking* e le discriminazioni - cioè quello che stiamo affrontando con l'attuazione della legge n. 77 - parla agli uomini. Se non sono gli uomini che in prima persona si assumono la responsabilità nei comportamenti individuali, nelle scelte politiche e nelle modalità con cui si relazionano, ovviamente il fenomeno necessiterà di tempi molto più lunghi per essere affrontato. Questo è un elemento di responsabilità. So che nella composizione della Commissione dovremo vedere la presenza di uomini; ogni partito

dare loro la possibilità di tornare in dimensioni di sicurezza nella propria vita affettiva e lavorativa. Questo aspetto riguarda il tema del lavoro delle donne, che non è escluso dall'attuazione della Convenzione di Istanbul. C'è poi un tema straordinariamente importante, quello della prevenzione. nel modo seguente: abbiamo avviato nella precedente legislatura linee guida sull'educazione al rispetto dell'integrità della persona all'interno del percorso formativo. Ma guardate che l'educazione al rispetto - si diceva all'affettività, che vuol dire rispetto dell'integrità delle persone - è un tema straordinariamente complesso e difficile: significa dire sia alle ragazze che ai ragazzi che nessuna e nessuno è proprietà di un altro; significa dire ai ragazzi che non si ama perché si possiede o perché si impedisce la libertà di un sì o di un no nei rapporti affettivi. Vuol dire anche dire alle ragazze che devono stare attente ai segnali nei rapporti affettivi

Questo significa tante cose anche nell'educazione degli adulti rispetto ai rapporti affettivi in famiglia. Ebbene, c'è una grandissima responsabilità sul terreno della prevenzione. Proprio su questo terreno dobbiamo sapere che la Convenzione di Istanbul parla a più soggetti: parla ai percorsi formativi sin dalla prima infanzia; ai percorsi che riguardano la comunicazione pubblica - se mi posso permettere - sia istituzionale sia dei *media*. Anche i linguaggi che si usano sono importanti da questo punto di vista per creare un contesto in cui

- stiamo violando un diritto umano e, quando si parla di diritti umani, la responsabilità pubblica, dello Stato e di tutte le sue articolazioni è un punto fondamentale. fondamentale. Veniva ricordato - lo dico anch'io - che siamo stati il primo Parlamento, la prima Nazione a ratificare la Convenzione di Istanbul; nessuno, però, dice più

dal punto di vista dello Stato, rispetto a tutto ciò che interviene discriminando le donne fino al femminicidio. C'è, cioè, una responsabilità diretta delle istituzioni pubbliche quindi, a partire dallo Stato centrale e da tutte le sue componenti governative - sul contrasto - come dice la legge - di ogni aspetto che esattamente discrimina e fa violenza sulle donne. Colleghi, questo è un punto importante perché, se c'è una responsabilità diretta,

*(L-SP-PSd'Az)*. Onorevole Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, a volte mi chiedo se fosse necessaria una parola nuova come femminicidio per indicare una situazione che è sempre esistita, ovvero la violenza sulle donne. Probabilmente e fortunatamente c'è stata un'evoluzione culturale e giuridica, sulla base della quale si è passati dal delitto d'onore, ancora realtà negli anni Settanta, all'attuale impianto normativo e all'attuale percezione dei fatti. L'ex neologismo «femminicidio» non è una parola in più sul vocabolario, solo se mostra un'inversione della prospettiva, e cioè la qualificazione di un atto di violenza sulla base non di chi sia la vittima, ma del motivo per cui è stato commesso. Mi spiego meglio: non c'è femminicidio quando la vittima è donna; c'è femminicidio quando la vittima è donna in quanto donna. Il fenomeno, oltre che essere studiato, deve essere soprattutto arginato. Fermo restando che il garantismo, parte fondante della nostra Costituzione e dogma per tutti coloro che in essa credono, inteso come il principio secondo il quale l'imputato non possa essere considerato colpevole fino a sentenza definitiva e secondo il quale la pena debba essere rieducativa, è un caposaldo, esso non può e non deve limitare le vittime.

analizzando i dati già in nostro possesso; il tutto volto al fine di dotare tutti i soggetti coinvolti di strumenti idonei e adeguati alla repressione del fenomeno. Se vogliamo parlare di prevenzione non possiamo rimanere sordi di fronte ai segnali d'allarme che le donne lanciano e che rimangono troppo spesso inascoltati. È frustrante, tutte le volte che leggiamo di un cosiddetto femminicidio, scoprire che sia stato preceduto da denunce e richieste d'aiuto rimaste inascoltate. È umiliante constatare che spesso si tratti di tragedie annunciate. È evidente, quindi, che le misure di prevenzione non siano sufficienti e che sia necessario intervenire per fornire alle Forze dell'ordine e alla magistratura strumenti più efficaci per proteggere quelle donne che hanno il coraggio di denunciare, ma anche quelle donne che, per vincoli culturali, economici o per paura, sono costrette a subire e a soffrire in silenzio. Va sostenuto l'accompagnamento delle donne vittime di violenza durante l'*iter* processuale, che spesso si ritorce contro le vittime stesse. Deve essere garantito l'anonimato e la riservatezza delle indagini e va potenziato il servizio dei centri e delle associazioni che operano sul territorio. Nel rispetto del caposaldo del liberalismo, secondo il quale la libertà di ogni uomo debba finire solo dove inizia quella di un altro, dobbiamo pensare a interventi organici, che consentano di proteggere le vittime prima che i loro carnefici. In Italia ci vogliono leggi chiare, difficilmente interpretabili, processi rapidi e pene certe. Pene certe: su questo mi vorrei soffermare. È grottesco ricordare che la fatica di tante donne che ha portato al riconoscimento del reato di *stalking* è stata vanificata dalla depenalizzazione improvvida di tanti reati minori ma ugualmente odiosi, con il cosiddetto decreto-legge svuota carceri. Vorrei soffermarmi sull'idea di interventi di carattere sociale, educativo e formativo. Questo tipo di reato, purtroppo, si può combattere non con il codice penale, ma con un'evoluzione culturale che deve iniziare nelle famiglie, che sono la prima forma di società naturale, e nelle scuole; scuole che devono essere non solo luogo di istruzione, ma anche di educazione delle prossime generazioni. Comunicando il voto favorevole di Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione all'istituzione della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, per tutti i sopracitati motivi, vorrei concludere ricordando a noi tutti le vere vittime innocenti, incolpevoli ma mai inconsapevoli, che attraversano queste tragedie famigliari come fantasmi silenziosi: i bambini. Il silenzio degli innocenti è ciò che più pesa sulle nostre coscienze e che io auspico costituisca l'impegno principale di questa Commissione. Una raccomandazione è rivolta a tutti noi: non perdiamo la possibilità di realizzare fatti concreti, perché rallentati da differenze ideologiche o di *background* culturale. Non rendiamoci protagonisti dell'ennesima occasione persa.

«femminicidio» suona molto male come parola, ma serve a definire in un modo appropriato la categoria criminologica del delitto perpetrato contro una donna; omicidio brutale di un essere umano, e in questo caso si ammazza non soltanto una donna, ma anche la sua famiglia e i suoi figli, che rimangono orfani: si vuole ammazzare, più o meno inconsciamente, il simbolo della continuità della vita. È necessario pronunciare questa parola per capire e spiegare meglio i contesti, per cercare di non banalizzare il fenomeno e soprattutto per non ridurlo - come a volte capita - quasi a una pura invenzione mediatica.

fenomeno non trova risoluzione e continua a perpetrarsi. Nel 2017 sono morte 113 donne, due di loro erano in attesa di un figlio, per lo più uccise da mariti, compagni o *ex* compagni, incapaci di accettare la fine della relazione o la volontà della *ex* compagna di ricostruirsi una vita al di fuori di lui. Oltre alle vittime, in prima linea non vanno dimenticati i bambini e i ragazzi, che in seguito a questi delitti si sono ritrovati orfani di madre, spesso col padre in galera, o di entrambi i genitori, nei casi di omicidio-suicidio. In Italia sono oltre 2.000 gli orfani del femminicidio. E a questo proposito voglio ricordare con grande orgoglio la battaglia di Forza Italia nella scorsa legislatura, quando nel disegno di legge per gli orfani dei femminicidi, grazie all'emendamento a prima firma dell'onorevole Carfagna,

Tra l'altro, Mara Carfagna è stata l'ultimo Ministro delle pari opportunità. Ai 60 ragazzi rimasti orfani nel 2017 se ne aggiungono circa 20 nei primi sei mesi del 2018. Essi, le vittime secondarie, hanno un'età che va dai cinque ai quattordici anni e la prospettiva di una vita molto difficile di fronte a loro. Ricordiamo l'ultimo caso di pochi giorni fa, quando un padre ha buttato la bambina di sei anni dal balcone, ferendo anche il fratello. Il femminicidio, anche se scoperto dai media e preso in considerazione dalla politica solo da qualche anno, non è certo un fenomeno di oggi. La violenza maschile sulle donne ha un carattere strutturale - come è stato detto - e non emergenziale, come ci ricorda appunto la Convenzione di Istanbul, che abbiamo ratificato la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa, detta Convenzione di Istanbul, ha permesso all'Italia di fare un ulteriore passo avanti nel contrasto di ogni forma di violenza, soprattutto nei confronti delle donne. Vi confesso di essere profondamente disgustata quando un capo religioso di qualche comunità, nel nostro Paese, ha il coraggio di affermare che è giusto picchiare una donna quando non ubbidisce.

fare una difesa a fasi alterne. Più volte ho avuto modo di ribadire con forza che la violenza nei confronti delle donne è un crimine contro l'umanità, che deve essere represso represso in ogni modo possibile. L'ho fatto in occasione della citata ratifica o nel 2009, quando convertimmo in legge, grazie al ministro Carfagna, ultimo vero Ministro delle pari opportunità, il decreto-legge del Governo Berlusconi sullo *stalking*.

l'ex ministro Boschi - ha deciso solo poco prima della scadenza elettorale di fare il piano antiviolenza, quello che aspettavamo da tre anni - senza dire una parola aveva infatti accettato, nel luglio del 2014, che non ci fosse più l'arresto

Ma da giugno, da quando si è insediato il nuovo Governo, ad oggi non ha detto una sola parola. Eppure, più di trenta donne e vari bambini sono stati uccisi. cento dei femminicidi è stato preceduto da una misura cautelare che disponeva il divieto di avvicinamento, ma purtroppo molte donne, nonostante tale divieto, hanno accettato l'ultimo appuntamento per loro fatale. Vi confesso che sono stata molto perplessa quando in Commissione è stato approvato l'emendamento per far sì che la Commissione duri soltanto un anno; poi però mi sono ricordata il grandissimo impegno e il lavoro che la precedente Commissione ha svolto in

Abbiamo sentito l'ANCI, la Conferenza Stato-Regioni, le associazioni di volontariato, i medici, il Garante dell'infanzia, il Capo della polizia, il Comandante dei carabinieri, il ministro Orlando - ne sapeva poco - l'Unione delle camere penali, il MIUR canali di informazione per dare un codice etico contro la spettacolarizzazione, che è sempre uno stimolo all'emulazione. Presentammo anche un questionario a tutte le procure sui procedimenti penali per la violenza di genere, ma solamente un terzo delle procure ha ad esso risposto. La cosa che emerge e che dovrà essere affrontata è che le procure non si parlano: ad esempio, il tribunale civile e il tribunale dei minori non si parlano e succede che, in casi di separazione con denuncia di violenza e maltrattamenti da parte della donna, il tribunale dei minori preveda l'affido condiviso. Ciò significa proprio che la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra. Mi auguro che queste criticità vengano affrontate dalla prossima Commissione. Noi certamente abbiamo il dovere morale di proseguire il percorso iniziato nella scorsa legislatura e mettere a nudo le criticità emerse. Certo, il più delle volte siffatti omicidi potrebbero forse essere fermati, ma sono tanti i casi in cui procure o Forze dell'ordine non hanno gli strumenti adeguati per fermare colui che poi sarà l'assassino. A questo punto, voglio fare un grande apprezzamento per il lavoro delle Forze dell'ordine: ho incontrato operatori sensibili e formati per raccogliere e sostenere le donne che avevano che avevano il coraggio di fare denuncia. Spero che nella prossima legge di bilancio, piuttosto che regalare soldi, il Governo decida di assicurare i giusti fondi per le Forze dell'ordine. *(Applausi

fa niente contro le bambine e che non si picchiano le donne neanche con un fiore. Forse qualche madre potrebbe cominciare a dire questo. Si è parlato della scuola, senatrice Fedeli. Sarebbe bene, senza inventarsi cose nuove, potenziare la settimana rosa contro la violenza che, per un protocollo d'intesa, i ministri Carfagna e Gelmini fecero, prevedendo che una settimana all'anno, in tutte le scuole dalle primarie alle superiori, si parlasse di tale tema. Ebbene, sono passati quasi dieci anni. Certo, la formazione culturale nel nostro Paese è molto giovane da questo punto di vista: è stato ricordato il diritto di famiglia del 1975, il delitto d'onore del 1985. Fino a trentasette anni fa il femminicidio nel nostro Paese era protetto dallo Stato, ed è stato ricordato come la violenza sessuale

Signor Presidente, devo fare una doverosa premessa. Io sono in Parlamento dal 2013 e vi posso assicurare che la lentezza del processo legislativo è una scusa:

che avete bisogno di cinque anni, significa che non avete alcuna intenzione di voler risolvere, arginare o provare almeno ad arginare il fenomeno. Significa che forse non si è consapevoli del fatto

ogni volta che si istituiva la Commissione di inchiesta. Volete qualche esempio? Per approvare la legge Fornero avete impiegato diciannove giorni; per il legittimo impedimento

concluso nella scorsa legislatura, perché non vogliamo perdere quel bagaglio di informazioni utili raccolte. Noi vogliamo dare continuità; vogliamo rafforzare e definire il percorso da intraprendere oggi seguendo tratti ben precisi. Innanzitutto, riteniamo che bisogna occuparsi fattivamente delle dimensioni del fenomeno femminicidio e violenza di genere in Italia. Occorre esaminare e perfezionare il quadro normativo in essere e la valutazione di impatto di alcuni profili delle norme stesse. La giurisprudenza sul tema dovrà essere più chiara, univoca e non interpretativa per permettere un'applicazione incisiva. Bisognerà incentivare il monitoraggio degli interventi di rete a tutela delle vittime e dei familiari; sostenere le azioni di protezione delle vittime e quelle di prevenzione del fenomeno; evidenziare ulteriori criticità, trasformandole in prospettive risolutive con adeguati atti legislativi. Queste sono alcune delle azioni che intendiamo porre in essere. C'è tanto da fare, molto da mettere in pratica, molto altro da fare. Le cronache quasi quotidianamente riportano racconti di omicidi, di violenze, di soprusi e di coercizioni, che spesso appaiono come il tragico epilogo di storie di sottocultura, di vite vissute all'insegna della brutalità, della violenza tossica o, peggio, della dipendenza, della sopraffazione, della prevaricazione dell'uno sull'altro. Non sempre, purtroppo, la violenza sulle donne e di genere esula dal concetto di ceto sociale e di benessere economico. Signori, da Nord a Sud, dall'illetterata alla laureata, dalla giovane all'anziana, indipendentemente dell'abitudine sessuale che la natura ci consegna, quando si parla di violenza si parla di un atto terribile, che può tradursi talvolta in vera e propria tragedia. Femminicidio, omofobia e bullismo sono atti e abusi che colpiscono tutti e per cui tutti dobbiamo sentirci responsabili. Di femminicidio e di violenza di genere muore una persona ogni tre giorni. Le statistiche parlano chiaro. Le percentuali risultano troppo alte per un Paese che si dice civile: nei primi sei mesi del 2018 sono state uccise già 44 donne, il 30 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Al contrario, il dato di chi sporge denuncia è molto basso, solo il 12 per cento di chi ha subito violenza e fra i reati più denunciati figurano lo *stalking* e la violenza domestica. Emerge anche il riscontro collegato alla non denuncia:

Un sistema di questo tipo certamente non consente tutela e spinge quindi a rimanere silenti di fronte alla violenza sia in ambito familiare che lavorativo. Il bilancio varia da Regione a Regione e le morti confermano il triste primato della Lombardia, con il numero più alto di donne assassinate, 11, seguita poi da Campania (6), Piemonte (5), Lazio (4) e Toscana (3). Due i casi di femminicidio registrati in Liguria, Veneto, Abruzzo e Calabria, mentre le restanti Puglia, Basilicata, Marche, Emilia-Romagna, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia-Giulia e Sicilia. È il caso dì È il caso dì Rossana, la giovane donna uccisa a Milano dal marito, quello che dopo il delitto è andato a giocare alle *slot machine*; è il caso di Sara, la ventiduenne romana, arsa viva in una strada della periferia di Roma dall'ex fidanzato che non accettava la fine della loro storia; è il caso di Federica, uccisa dal marito proprio il giorno in cui avrebbe dovuto formalizzare l'atto di separazione; è il caso di Elisabeth, strangolata davanti ai suoi figli dal convivente, reo confesso; è il caso di Noemi, la sedicenne della provincia di Lecce seppellita ancora viva nonostante le coltellate inferte dal suo aguzzino, il cui giovane fidanzato è stato condannato (con futuri premi e sconti annessi e connessi dall'attuale legislazione) a soli 18 anni ed 8 mesi di detenzione proprio pochi giorni fa; è il caso dì Vincenzo, attivista *gay*, ucciso ad Aversa, dal fidanzato di una sua amica *trans* per gelosia; è il caso di Fernanda, 77 anni, trovata in casa con un laccio intorno al collo e legata al termosifone, uccisa dal vicino di casa con cui aveva una relazione, che lui voleva rimanesse segreta. E si potrebbe continuare a lungo in un drammatico elenco di storie che, per quanto siano numerose e spesso sovrapponibili, diventerebbero tristemente asettici numeri e fredde statistiche, facendoci allontanare dal fulcro principale: fermare questa orribile mattanza che sembra senza fine, per cui abbiamo l'obbligo di dire basta! Nella precedente legislatura il Governo ha legiferato, con il decreto-legge n. 93, ad agosto del 2013, e successive modificazioni con la Legge 119, nell'ottobre 2013, per il contrasto della violenza di genere con l'obiettivo di prevenire il femminicidio e proteggere le vittime. Come era prevedibile, quella legge non ha dato i risultati sperati. Fanno fede i dati del Ministero dell'interno che sono impressionanti: negli ultimi cinque anni si registrano una media di 160 omicidi all'anno, ciò significa che ogni due giorni in Italia viene uccisa una persona dal proprio *partner*. Perché? Perché, purtroppo, di fatto, l'intervento legislativo prevede solo una forma di tutela *ex post*, ad omicidio già commesso. A nostro avviso il legislatore dovrebbe intervenire preventivamente, con maggiore, efficacia, incentivando la cultura dell'educazione, volta ad arginare siffatti fenomeni ed a tutelare maggiormente tutte quelle persone che invano denunciano episodi di violenza domestica posti in essere dalle stesse persone, per mano delle quali, poi, verranno uccise. Non dimentichiamo poi che la violenza di genere provoca vittime anche tra chi resta, un dramma nel dramma. Circa il 70 per cento dei figli di coppie artefici di episodi di violenza, avrebbe assistito all'atto ed è stato stimato che dal 2000 ai giorni nostri vi è un alto numero di orfani di femminicidio, circa 500 nel corso

un fatto che purtroppo accade troppo ripetutamente e che inquina la società civile, la convivenza, la cultura del vivere mondiale, i diritti umani: è un fatto che bisogna debellare, affamare. Colleghi, abbiamo il dovere di assolvere all'obbligazione di assicurare la protezione dei diritti fondamentali, sia *de iure* che *de facto*. "Quante donne sopraffatte e dal peso della vita e dal dramma della violenza, il signore le

È del 12 ottobre la notizia apparsa su ANSA che leggo testualmente: un presunto *stalker* può essere trattato come un presunto mafioso e gli può essere applicata la misura di sorveglianza speciale per la pericolosità sociale anche da imputato

Paola Di Nicola: "Il femminicidio ha la stessa valenza sociale e culturale della mafia. Si deve pretendere dallo Stato lo stesso sforzo che si impiegherà a combattere il fenomeno mafioso perché il femminicidio, inteso in senso ampio, arriva ad ammazzare, nel disinteresse assoluto, più della mafia, uccide la vita e la dignità di intere

che se ne debbano fare altre, tante, insieme, perché l'attenzione va cambiata, il contesto va ripensato, l'elaborazione delle proprie emozioni può essere un cammino lunghissimo, inedito, in un percorso di assunzione di responsabilità che veda impegno, consapevolezza e volontà,

Signor Presidente, le chiedo di farsi portatore presso il Governo della richiesta di venire a riferire in quest'Aula sulla vicenda del TAP in Puglia e quindi sulla prevista riapertura dei cantieri nel Comune di Melendugno. Sappiamo infatti di una riunione svoltasi ieri a Palazzo Chigi, convocata dal presidente Conte, alla quale hanno partecipato i ministri Costa e Lezzi e alla quale è stato concesso di partecipare - cosa singolare ed irrituale solo ai deputati e consiglieri regionali pugliesi del MoVimento 5 Stelle, oltre che al sindaco di Melendugno. Alla conclusione di questo incontro, la ministra Lezzi, che fino a qualche mese fa ha girato in lungo e in largo il Salento facendo incetta di voti, dicendo che avrebbe revocato il progetto in quindici giorni, ha detto

Sono le dichiarazioni del sindaco di Melendugno, riportate dalle agenzie di stampa, ma anche in un *post* pubblico sul profilo dello stesso, secondo le quali il sindaco avrebbe affermato come gli sia parso che il *premier* Conte richiedesse soccorso alla procura, così da toglierlo dall'angolo in cui si trova. Credo che queste siano dichiarazioni molto gravi e necessitino di un chiarimento urgente da parte del *premier* Conte in Aula e per questo le chiedo di sostenere la mia richiesta.

trucidato all'interno del consolato saudita di Ankara, consolato nel quale l'uomo si era recato per sbrigare delle pratiche per il suo imminente matrimonio. Come già fatto l'11 ottobre dai senatori della Commissione esteri del MoVimento 5 Stelle, vorrei ricordare, semmai ce ne fosse bisogno, che le torture e lo smembramento del corpo contravvengono a tutte le regole diplomatiche, ma ancor di più a quelle morali e civili della comunità internazionale. La colpa del giornalista è stata quella di aver criticato l'operato della famiglia reale e, in particolare, il principe ereditario Mohammad bin Salman Al Sa'ud. Pensate, quest'ultimo, secondo la propaganda saudita, sarebbe un innovatore e un moderato che, però, a quanto pare, non tollera i giornalisti. Tale orrore potrebbe avere spazio in una puntata dei «Soprano», invece i mandanti appartengono ad una famiglia ancor più brutale, quella saudita, cui però buona parte dei Paesi del mondo hanno relazioni economiche, in particolari gli Stati Uniti, dove l'ultimo ordine di armi dei sauditi ammonta a ben 110 miliardi di dollari, di cui 15 già versati. Eppure, anche negli Usa questa volta c'è molto imbarazzo nel difendere l'alleato. Dobbiamo pretendere chiarezza su questo atto mostruoso e condannare chi lo ha compiuto con la stessa fermezza con cui in passato questo Parlamento ha ha condannato episodi simili. Concludendo, a questa dittatura i precedenti Governi hanno permesso la vendita di armi prodotte in Sardegna, violando la legge n. 185 del 1990 che, a questo punto, è necessario riformulare in forma restrittiva. Mi dedicherò

Signor Presidente, onorevoli colleghi, da troppi anni una categoria di dipendenti pubblici è vittima di riforme tanto attese e desiderate, ma mai realizzate. Mi riferisco al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La carenza di organico dei Vigili del fuoco è ormai cronica e, insieme alla loro età media avanzata, causa un problema di sicurezza sul lavoro che potrebbe pregiudicare l'efficienza dei soccorsi. Colleghi, è necessario fare tesoro delle emergenze vissute nel nostro Paese, quali terremoti, alluvioni e crolli. Tali esperienze confermano la necessità di adeguare il Corpo dei vigili del fuoco alle esigenze del Paese, anche attraverso le assunzioni di quei precari che operano da anni in attesa di essere stabilizzati, come tutti coloro che, per età non adatta a ricoprire un ruolo operativo, potrebbero essere impiegati per colmare le carenze di personale logistico organizzativo. Una delle mancate riforme da parte dei Governi precedenti, che reputo immorale nei confronti di chi giornalmente rischia la propria vita per salvare quella altrui, è la mancata equiparazione dei ruoli, delle qualifiche e delle retribuzioni a quelle delle Forze di polizia. Non è pensabile infatti che appartenendo allo stesso Ministero dell'interno, i Vigili del fuoco percepiscano trattamenti retributivi notevolmente inferiori alle altre Forze dell'ordine. Considerato che il Governo con il decreto sicurezza ha stanziato notevoli risorse, chiedo allo stesso che gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco vedano riconosciuti i loro diritti e meriti e possano finalmente svolgere efficientemente il loro inestimabile lavoro,

La nostra delegazione è stata eletta tardivamente. Per la prima volta dal 1949 è decaduta la delegazione precedente, cioè per la prima volta l'Italia non aveva alcun rappresentante e ciò non era mai successo. Non essendo ancora stata convocata la delegazione congiunta di Camera e Senato e non avendo ancora eletto un Presidente, non abbiamo potuto partecipare, non noi ma tutta l'Italia, il Paese, a nessuna delle Commissioni che fanno parte del Consiglio d'Europa. Credo che questo sia un problema serio, quindi, siccome sono i Presidenti di Camera e Senato che devono convocare la delegazione, chiedo ufficialmente che venga fatto al più presto e lo faccio veramente senza nessuno